La seduta è aperta

estrema e che avrei voluto evidenziare ieri se non fossi stato io a presiedere. Nel corso delle precedenti dimissioni - perché ormai abbiamo questa tradizione del voto sulle dimissioni - gli interessati hanno sempre sollecitato un voto a sostegno delle proprie dimissioni. È legittimo che vengano presentate e portate avanti. Ieri l'ex collega Vernetti chiese a me e, per mio tramite, al mio Gruppo di votare respingendo le proprie dimissioni.

a stabilire finalmente una giornata in cui si possono discutere tutte le eventuali, residue, dimissioni in modo da capire se questa è una prassi

ringrazio, senatore Calderoli, per la serietà e la fermezza con cui ieri ha presieduto l'Aula. Ha ritenuto, giustamente, con il suo giudizio politico, di fare quel giro di osservazioni, ma le regole sono state rispettate.

ormai estremamente urgente e che ho fatto presente ieri al presidente Calderoli, il quale è stato molto cortese nel fornirci alcune informazioni; altre informazioni riferite (non certo per responsabilità del presidente Calderoli, che non poteva saperle) non risultano però conformi a ciò che ci è stato detto. Mi sto riferendo, signor Presidente, alla questione che riguarda i vitalizi dei parlamentari, a lei ben nota perché ella ha ricevuto un articolato abbastanza

che venga posta a conoscenza dei parlamentari. Ad ella, però, che è stato così sensibile all'attività di questa Camera alta e dei singoli senatori, non potrà sfuggire il fatto che una materia così delicata, che è stata oggetto di una lunghissima campagna di stampa

visto che alla fine dell'anno probabilmente coloro che oggi hanno 57 anni dovranno maturare altri tre anni di lavoro per andare in pensione. Signor Presidente, sarebbe cosa buona ed estremamente opportuna che i colleghi senatori venissero a conoscenza dell'articolato che verrà posto alla discussione del Consiglio di Presidenza prima che esso possa

il numero delle persone che compongono il Consiglio di Presidenza e che adottano questa deliberazione e i soggetti su cui ricade la deliberazione stessa. Ora, siccome probabilmente l'estrema articolazione della proposta inviata il 16 maggio ha reso difficile fornire una risposta a coloro che l'hanno inviata, penso di poter sommessamente richiamare la sua attenzione affinché la deliberazione del Consiglio di Presidenza avvenga dopo che i Capigruppo abbiano ricevuto il testo articolato, che a ieri pomeriggio non mi risulta sia stato loro consegnato (forse

Voglio assolutamente rassicurarla. Naturalmente le competenze sono del Consiglio di Presidenza, ma almeno per quanto riguarda la mia visione di tali questioni non mi ha mai sfiorato l'idea - per questo la rassicuro

situazione che si è venuta a creare. Vorrei ribadire, anche perché sono membro della Giunta, che ieri in quest'Aula si è verificata una situazione assai grave di incompatibilità, che non può essere misurata a minuti, né a ore, né a mesi, ma che è incompatibile e quindi, tautologicamente, non dovrebbe mai esistere: mai esistere: un senatore, seppure per pochi minuti, ha rappresentato due collegi, la Puglia e il Piemonte. È una situazione di incompatibilità che non dovrebbe sussistere mai che non è risolvibile solo perché dopo cinque minuti il senatore opta. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che, bisogna dirlo, su questa decisione della Giunta si è ritrovata compattamente tutta la opposizione e parte della maggioranza, e questo mi preoccupa molto perché, ripeto, sono situazioni di incompatibilità che non dovrebbero mai sussistere e che quindi credo debbano essere risolte anche regolarmente in quanto, ripeto, è impossibile, sia pure per un minuto, che un senatore possa rappresentare in Senato contemporaneamente due collegi. lei pone due questioni con la pacatezza e la serietà che sempre la contraddistinguono. Sulla prima questione,

senatore Di Lello Finuoli, la Giunta è composta da senatori di uno schieramento e dell'altro e credo non

Governo - che, per una scadenza prevista dal decreto-legge convertito in legge sulle missioni internazionali, entro il 30 giugno il Governo avrebbe dovuto riferire alle Commissioni competenti, cioè e difesa, di entrambi i rami del Parlamento su ciascuna delle 17 missioni menzionate in quel decreto. Mi risulta da agenzie di stampa che il Governo abbia relazionato su una missione in una

notizie in merito. Una scadenza e un impegno previsti dalla legge e votati, tra l'altro, con pochissimi voti contrari alla Camera e confermati all'unanimità qui al Senato;

Vede, senatore, questo secondo me non allude al fatto che ci sia stata una violenza; nessuna violenza sul senatore Vernetti. Forse allude ad altro: il senatore Vernetti non ha, nella sede propria, affermato con dignità e con coraggio il proprio punto di vista e ha preferito lavorare nell'ombra tradendo la fiducia che lo lega a questa maggioranza e agli impegni che aveva assunto.

Lo è perché, non essendo prevista la necessità di operare l'opzione entro un termine certo, ed essendo il sistema un sistema che spinge verso le candidature multiple, la possibilità di una contemporanea elezione in diversi collegi - a prescindere dal fatto che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione e non il singolo collegio, come stabilisce la Costituzione si può produrre in ogni momento, e nel momento della prima verifica dei risultati degli eletti e successivamente. Se noi quindi ci poniamo di fronte a tale questione

terza questione - è che, come risulta anche dai giornali e dalle agenzie di ieri, i componenti del Gruppo dell'Ulivo al Senato si sono divisi nella decisione, a dimostrazione fatto che non c'è stata alcuna pressione della Presidenza perché il Gruppo dell'Ulivo si comportasse in un modo piuttosto che in un altro, e che quindi ciascuno è stato ritenuto e garantito libero nella propria decisione.

che non c'è stata alcuna preordinazione della decisione della Giunta con una precostituzione della posizione del Gruppo dell'Ulivo. Queste erano le questioni che volevo affrontare ringrazio i colleghi perché mi pare che i toni del dibattito odierno, e anche la sua decisione, Presidente, assunta poc'anzi su sollecitazione del senatore Calderoli, siano adeguati alla delicatezza della questione. Colleghi, ho ritenuto, dopo l'intervento del senatore Calderoli, che anche i toni forti della chiusura della seduta di ieri imponessero un minimo di chiarimento, che stiamo facendo.

rispetto all'obbligo del Governo di venire a riferire sullo stato di avanzamento delle missioni militari all'estero. Anche noi sosteniamo questa urgenza, anche per avere un aggiornamento pronto sugli esiti della Conferenza sulla giustizia in Afghanistan che fa parte di questo pacchetto di note. Volevo altresì dire che in Commissione esteri abbiamo già sollevato la questione, quindi aspettiamo che il Governo sia convocato in maniera rapida.

la prima questione che volevo rimanesse a verbale è quella che ella ha sollevato quando, rispondendo alla collega Finocchiaro, faceva notare come ogni valutazione in merito ai comportamenti del senatore Vernetti sia quanto meno ingenerosa in questa sede, visto

esercitare quel diritto al contraddittorio e al confronto che è una regola minima di qualunque democrazia, anche di quelle di origini sovietiche, ormai obsolete ed in disuso. Quindi, fermo restando che le perplessità in merito a quanto è successo ieri sul caso Vernetti si colgono soltanto analizzando i numeri, perché dalla loro verifica probabilmente possono essere considerate condivisibili le riprovazioni delle trame singole, signor Presidente, restano ancora più criticabili le trame complesse, quelle ordite con sottili messaggi, indicazioni e passaggi che costringono molti, inconsapevolmente, ad essere soggetti di un gioco molto più grande. Alla fin fine, Vernetti esercitava un diritto all'autodifesa che oggi gli viene negato in quest'Aula, per cui era legittimato anche a mettere in campo comportamenti non molto in linea; per la verità, è molto più complicata la situazione di coloro che, invece, quelle trame hanno avuto il coraggio di ordire. Sono inoltre d'accordo con la collega

capacità di interpretazioni diverse, di contrapposizione, di utile percorso costruttivo nell'evolversi di una decisione), poiché in questo caso non è così: il problema serio era, infatti, che non esiste nessuna norma,

in Giunta c'è stato il contraddittorio; un contraddittorio relativo, però, perché ci sono stati coloro che hanno espresso le proprie opinioni e coloro che si sono dovuti accodare alle opinioni altrui. Questa è stata la grande differenza ieri: ieri: chi non aveva ricevuto nessun tipo di indicazione e chi invece aveva ricevuto l'indicazione di accodarsi. Signor Presidente,l'istituto dell'autodichia, che dovrebbe garantire l'indipendenza del Senato e che consente al Senato di operare valutazioni pure in merito alla sua composizione e quindi alla legittimità delle elezioni, dovrebbe vedere un uso più equilibrato, perché si tratta di un potere che deve costituire una garanzia di correttezza e di indipendenza; in questo momento, purtroppo, viene esercitato dal Senato come un potere che deve garantire soltanto una cosa: la prepotenza, contro la quale mi batterò Non voglio fare il pignolo, ma un senatore in qualsiasi Giunta o Commissione ha il diritto di esprimere quello che vuole, quando lo ritiene,

Onorevole Presidente, sono convinto di quanto ha detto la senatrice Finocchiaro. Non c'è stata pressione da parte dei Presidenti di Gruppo verso i colleghi. Ho troppo rispetto dei colleghi Presidenti di Gruppo per ritenerlo. C'è stata un'indicazione di voto da parte del Gruppo. Non ho nessuna preoccupazione ad affermare che ieri l'indicazione di Gruppo di Alleanza Nazionale relativa alle dimissioni del senatore Vernetti era di votare contro. Nel segreto dell'urna, non posso garantire per tutti i 41 senatori del mio Gruppo, ma certamente l'indicazione era di votare contro le dimissioni del senatore Vernetti. Tuttavia, non è questo il problema. lo abbiamo sollevato ieri - prima il senatore Pera e poi, molto più modestamente, il sottoscritto - non partecipando al dibattito sulle dimissioni. sulle dimissioni. È vero ciò che ha detto il senatore Calderoli: credo che nessuno in quest'Aula possa negare che il senatore Vernetti non volesse lasciare il seggio di senatore.

il Governo in qualche modo incide sulla composizione di quest'Aula. Questo non è giusto, è scorretto,

viene eletto per volontà popolare; la volontà popolare aveva portato Vernetti in quest'Aula e il Governo gli ha imposto di dimettersi per fare il Sottosegretario. Pertanto, dal momento che ci sono ancora dimissioni in corso, rivolgo rivolgo lo stesso appello - forse inascoltato - che ho rivolto ieri: invito i senatori che ricoprono cariche di Governo e che hanno rassegnato le dimissioni a ritirarle e a riflettere. Se vogliono presentarle, lo devono fare liberamente e non perché c'è un'imposizione del Governo, una *condicio sine qua non* per continuare a far parte, da Sottosegretari o da Ministri, dell'attuale Governo. Questo è il ragionamento che dobbiamo fare in maniera molto chiara, lineare e forse anche pragmatica. Sulle

Un membro del Governo presenta le dimissioni perché il Governo gli chiede di farlo e perché, essendo i numeri in quest'Aula molto ballerini e molto fragili per la maggioranza ed essendovi una maggioranza

chiaro che venivano date, ma non sul serio! Come credete abbiamo fatto noi ad avere la maggioranza in tutte le occasioni nelle quali abbiamo respinto le dimissioni di membri del Governo? Perché voi avete votato contro le indicazioni del vostro Governo e vi siete dissociati dalla vostra maggioranza, una volta un Gruppo, una volta un altro, un'altra volta un altro ancora. Non è andata così? Non è questo il problema politico della vostra ipocrisia? PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, per favore.

e inopinatamente, invece, è stato sfortunato, perché nella maggioranza è prevalsa in molti

non vi è stata una tesi ragionevole ed una irragionevole e assurda. Vi erano due tesi a confronto, tra l'altro su un problema che si è posto in maniera rilevante proprio in ragione del fatto che la pluralità delle candidature ha determinato la questione della sussistenza o non del diritto di opzione, in capo a chi non aveva potuto esercitarlo al momento delle elezioni, ma si trovava poi in una situazione di possibilità prima sconosciuta. Sarà opinabile, discutibile, ma è una tesi che ha dei fondamenti seri e solidi,

un anno fa da parte di componenti del Senato potevano ritenersi politicamente sostenute dalla necessità di consentire al Senato una piena funzionalità di sostegno al Governo (perché si immaginava che i Ministri e i Sottosegretari non avrebbero potuto sostenere costantemente l'azione di Governo dovendo svolgere il loro ruolo nell'Esecutivo) dopo un anno e più credo che questa necessità sia venuta meno. Vi sono Sottosegretari che hanno partecipato costantemente ai lavori dell'Assemblea del Senato, Ministri che hanno partecipato costantemente ai lavori del Senato, tra i quali, oltre al ministro Turco qui presente, il ministro Mastella, che ha una responsabilità di grande peso: la loro doppia veste non ha certamente influito sulla funzionalità del Senato e sulla tenuta della maggioranza. Quando la maggioranza è andata sotto, sotto, è stata battuta per altre ragioni, politiche o magari di contingenza numerica, certamente non collegate alla presenza di senatori tra i banchi del Governo. il punto è allora un altro ed è questo il dato politico: in realtà, sul presupposto di tali dimissioni, nel campo del centro-sinistra si sono operate delle collocazioni precise, si sono assunti degli impegni, si sono fatte delle promesse, si sono date garanzie che Tizio sarebbe entrato a far parte dell'Assemblea del Senato perché Caio aveva presentato le dimissioni e queste sarebbero state accettate. Ieri, con l'accettazione delle dimissioni del collega Vernetti, certi impegni sono stati in parte disattesi. Qualcuno aveva garantito che la Giunta avrebbe assunto una certa decisione

di problema interno al centro-sinistra, che deve su di esso fare una riflessione. Ben venga la giornata dedicata alle dimissioni, perché non è possibile contrabbandare la volontarietà delle dimissioni quando invece, alla base, vi è una sostanziale redistribuzione delle funzioni e dei ruoli (per non dire delle poltrone) che in questo momento per l'Unione e per il centro-sinistra è particolarmente rilevante. Infatti, il centro-sinistra si è frazionato e non è un caso che ci sia stata una rottura e una polemica da parte di componenti già dei DS che non sono confluiti nel Partito Democratico, o di una parte del Partito Democratico, in polemica, però, nei confronti di questo nuovo soggetto. Signor Presidente, il problema è dunque tutto interno al centro-sinistra. Aggiungo che se il centro-destra non avesse partecipato alla votazione comunque la scelta della Giunta sarebbe stata quella che poi è risultata vincente, perché nel centro-sinistra la maggioranza ha votato in tal senso. Quindi non ci sono inciuci o trame particolari: vi è solo una scelta giuridica che ha sconvolto i piani dell'Unione.

Ascoltato quanto è stato detto prima, vorrei dire che la volontarietà delle mie dimissioni è totale e assoluta. Posso affermare di non essere stato pressato da nessuno a presentare le dimissioni. Anzi, Presidente, e la prego lei sa che intendo avanzare una sola richiesta, che ho ribadito anche ieri sera: che non passi troppo tempo perché le mie dimissioni vengano di nuovo calendarizzate in Aula.

questo atto. Ciò non è avvenuto, ma la prego, per cortesia, di non andare oltre i primi giorni della prossima settimana perché tale atto venga calendarizzato. Non posso più sopportare, onorevole Presidente, di essere impiccato ancora - non dico crocifisso, perché sarebbe troppo nobile - ad un atto che viene definito come l'espressione tipica (che tocca anche il Parlamento nel suo complesso) dell'arroganza del potere. Sono stato invitato da più parti a ritirare le dimissioni; ringrazio coloro che mi hanno rivolto tale preghiera, ma ho bisogno di parlare in quest'Aula perché i fatti siano chiari. Sono indifferente alle decisioni, comprese quelle che potrei prendere io; in questo momento sono interessato soltanto alla discussione della lettera che io, signor Presidente (e le motivazioni in parte le conosce), ho sottoposto alla sua attenzione. **Sul

ad un dibattito importante per la sua vita, ma credo poco seguito dall'opinione pubblica, un altro giorno di cattività si apre per padre Bossi. Mi appello alla sua sensibilità perché possa il Senato, al più presto, colmare una lacuna che è del Governo. Stamani, recandomi al Senato, signor Presidente, e passando davanti al Campidoglio, non ho visto gigantografie di rapiti, come mi è capitato di vedere in altre occasioni. *(Applausi Stamani, seguendo i telegiornali del mattino, non mi è capitato di vedere, come in altre occasioni, titoli di apertura che riguardavano i nostri sequestrati.

Non vorrei che un'istituzione che per definizione non può essere relativista, perché un'istituzione per definizione incarna i sentimenti e le relazioni che vive un Paese, non trattasse questo argomento alla stessa maniera e con lo stesso impegno. Non vorrei che il Paese cosiddetto reale ci avesse ancora una volta superati; ieri sera in piazza Santi Apostoli, su iniziativa di Magdi Allam, la gente si è riunita, a migliaia, contro la persecuzione dei cristiani nel mondo. La gente si è riunita, a migliaia, e ha fatto quadrato contro il relativismo che prende tutti quanti, contro l'apatia. Credo che il rischio maggiore che corriamo è quello dell'indifferenza. Forse tanti sequestri ci possono abituare ai sequestri;

Se fosse possibile nella serata - oggi c'è seduta - avere durante lo svolgimento delle interrogazioni la presenza del Governo che risponda in merito, lo comunicheremo in corso di giornata all'Aula. Faremo di tutto.

l'opposizione può chiedere, su iniziative che vengono dall'opposizione, magari non finite o non discusse in Assemblea, che ogni due mesi nella Conferenza dei Capigruppo si decida di affrontare qualcuna di tali questioni.

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge del senatore Castelli e di altri senatori della Lega contiene una delega al Governo per la nomina elettiva dei giudici di pace. Questa possibilità è prevista dalla nostra Costituzione, la quale, al secondo comma dell'articolo 106, ammette la possibilità di magistrati onorari di nomina anche elettiva.

come sicuramente il ministro Mastella starà confermando in questo momento al presidente Marini e al dottor Malaschini, e ha avuto un esito positivo dal punto di vista della capacità di rendere una giustizia vicina ai cittadini. Il ministro Mastella converrà altresì sul fatto che il valore - ancorché possa essere ridotto - delle controversie sottoposte all'attenzione del giudice di pace non per questo è meno rilevante,

per un senso della giustizia che si proclama non essere stato soddisfatto, quindi per il senso di offesa nei confronti della violazione della giustizia.

Nel nostro sistema, infatti, abbiamo avuto e ancora abbiamo qualche difficoltà (pur, lo ripeto, riconoscendo l'esito molto positivo di nell'individuare le caratteristiche e le modalità di reclutamento di questi soggetti. Il disegno di legge fatto proprio dal senatore Castelli individua alcuni requisiti, alcuni criteri necessari e propone di sciogliere il nodo attraverso un meccanismo elettivo nell'ambito di ciascun distretto di corte d'appello. È anche evidente, d'altra parte, che questa tematica sarebbe assolutamente innovativa per l'ordinamento giuridico italiano e richiede, quindi,

di rinviare la discussione o deliberazione su un determinato argomento ed io credo che questo rinvio possa essere ragionevolmente determinato in modo tale da riprendere la discussione in Aula del disegno di legge Castelli dopo aver affrontato le questioni di merito che la proposta pone nell'ambito della Commissione giustizia,

di esaminare attentamente il disegno di legge e anche, se possibile, di collocarlo su uno sfondo più ampio che può riguardare l'applicazione dell'articolo 106 della Costituzione repubblicana, un articolo assai importante per molti anni negletto. Interviene, però, un ulteriore e determinante motivo che mi induce a presentare la questione sospensiva.

nel suo insieme, che utilizza la copertura a legislazione vigente della legge per l'istituzione dei giudici di pace. Perciò, in una riunione della Commissione bilancio, il relatore senatore Albonetti ha sottolineato l'opportunità di acquisire conferma dal Governo sull'assenza dei profili finanziari relativi al testo in discussione che avrebbero dovuto determinare un parere della Commissione bilancio. Il sottosegretario Antonangelo Casula, che era che era presente alla riunione della Commissione bilancio in rappresentanza del Governo, ha rilevato che i criteri direttivi indicati nel provvedimento sono suscettibili di determinare oneri finanziari per il bilancio dello Stato; anche da parte del rappresentante del Governo è venuta la conferma della necessità di un'opportuna verifica sul disegno di legge nel suo insieme da compiere nell'ambito della Commissione bilancio e che non è stata compiuta. Anche per questa ragione, che è a mio giudizio determinante, noi chiediamo una sospensione della discussione di questo disegno di legge per poterne esaminare i profili finanziari e per poter dare luogo ad un confronto serio e approfondito nell'ambito della Commissione giustizia. *(Applausi dei

ma poi anche di natura formale legata, invece, ai rapporti tra maggioranza e opposizione. Intanto dico che *ictu* *oculi*, vista la composizione dell'Aula, sarà difficile opporsi a questa proposta, stante i i rapporti di forza che in questo momento vengono espressi. Questo, comunque, lo dirò alla fine. Dal punto di vista sostanziale lasciatemi esprimere soddisfazione per il fatto che ancora una volta - non credo sia la prima, sicuramente non sarà l'ultima è la Lega Nord a porre questioni che non sono mai state sollevate né nel Parlamento né nell'opinione pubblica. Mi correggano i colleghi se sbaglio, ma credo che sia assolutamente la prima volta che si tratta questa materia, che peraltro è prevista dalla Costituzione, in un'Aula parlamentare. Perché accade questo? È successo più volte in questi anni di Repubblica. I nostri Padri costituzionali hanno cercato di costruire, anche per quanto riguarda la giustizia, un sistema equilibrato, un sistema che ha dato alla magistratura, come è giusto che sia, un'amplissima autonomia e indipendenza, ma non si sono fermati a questo. Ho avuto per anni il piacere di vedere i magistrati sventolare la Costituzione di fronte a me quando intervenivo in svariate occasioni, anche solenni. Io li ho sempre invitati a leggerla tutta la Costituzione e non soltanto i pezzi che a ciascuno fanno comodo. Se leggiamo il Titolo IV, possiamo vedere, almeno a mio parere, che i nostri costituzionalisti hanno inteso, da un lato, dare appunto grandissima autonomia e indipendenza alla magistratura, così come vuole Montesquieu e come vogliono i princìpi delle democrazie sulle quali noi ci basiamo oggi, ma dall'altro hanno anche inteso introdurre dei princìpi per i quali il magistrato non diventasse una sorta di monade leibniziana senza

che recita: «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Questa frase è stata talmente dimenticata che, quando l'abbiamo reintrodotta nella scorsa legislatura, c'è stata una sollevazione da parte di molti magistrati che non capivano quale fosse il significato profondo di questa frase; qualcuno addirittura ha ironizzato dicendo: «Mah, sarà il popolo padano», non capendo che invece questa frase indica il fatto che il magistrato, quando giudica, non deve mai dimenticare non soltanto le leggi, non soltanto la dottrina ma che, come voi mi insegnate, fa giurisprudenza e quindi, giudicando ed emettendo sentenze, deve anche tener conto

fa giurisprudenza e di fatto, poi, in qualche modo legifera, perché se ne deve tener conto e spesso anche il Parlamento si adegua alle sentenze emesse dalla magistratura: spesso la magistratura anticipa le leggi che poi il Parlamento deve fare adeguandosi alla società che si evolve.

ma sono coloro che amministrano quella giustizia che spesso è la più spicciola, la più vicina al cittadino, che vuole giustizia non soltanto sulle grandi transazioni societarie o, purtroppo,

dei nostri Padri costituzionalisti sul tema: la famosa giustizia sotto l'albero, che è quella che poi serve a far sì che il cittadino abbia fiducia nello Stato e che purtroppo oggi non c'è,

per quanto riguarda appunto l'erogazione del servizio giustizia; oggi, senza giudici di pace, il servizio giustizia crollerebbe. Soltanto in materia civile (che è proprio il caso a cui facevo riferimento) all'anno: pensate, 1.200.000 cause all'anno! Una cifra gigantesca, che ormai ha superato in termini quantitativi il numero di cause portate a termine

non si può così, *ex abrupto*, approvare una norma di questo genere, che è totalmente innovativa, non soltanto dal punto di vista organizzativo, ma credo soprattutto dal punto di vista culturale; ma, colleghi, vogliamo andare avanti, vogliamo applicare questa norma, che credo potrebbe essere veramente positiva per il Paese? Vogliamo superare le paure ideologiche e culturali che ci attanagliano ogni volta che si vuole fare una riforma seria?

non creda lo si sia fatto soltanto per ragioni formali. Ora, mi perdoni il collega Brutti, ma con la questione sospensiva di fatto si vanifica il diritto dell'opposizione di discutere, perché non riusciamo neanche a fare la discussione generale;

e di fatto il diritto dell'opposizione di vedere non certo approvati ma esaminati approfonditamente i disegni di legge che propone viene vanificato. Credo che questo sia un tema sul quale, signor

dopo aver ottenuto dalla Presidenza la possibilità di esaminare il testo - in quanto inizialmente era stato considerato soltanto ordinamentale, mentre nella riunione di ieri della Commissione bilancio avevamo indicato invece la possibilità che il disegno

che il disegno di legge, prevedendo un'elezione diretta e generale, ha in sé dei costi palesemente riscontrabili.

ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Questo è uno dei motivi che mi inducono a chiedere al senatore Castelli di concordare sulla proposta avanzata dal relatore di un rinvio in Commissione, anche per poter eventualmente proporre profili di copertura corretti che possano determinare un assenso della Commissione

accennato in coda al suo intervento dal presidente Castelli. È evidente che le questioni incidentali le questioni incidentali fanno parte del procedimento legislativo e possono essere poste secondo le norme previste dal Regolamento; ma è altrettanto chiaro - e al riguardo bisognerebbe approfondire la riflessione che nei Regolamenti parlamentari certe norme, introdotte per consentire da parte dell'opposizione la discussione di proprie proposte, sono nate a seguito dell'introduzione, nel nostro sistema politico, e in parte nel nostro ordinamento costituzionale, di princìpi di natura maggioritaria, e che si è voluto, attraverso norme che si definiscono, più in generale, come statuto delle opposizioni (e che in qualche misura andrebbero meglio precisate anche sul piano costituzionale), offrire garanzie all'opposizione affinché le sue proposte possano essere discusse in modo approfondito ed eventualmente approvate o respinte con la stessa attenzione, intensità e dignità con cui vengono trattate le proposte provenienti dalla maggioranza o dal Governo, senza alcuna

sono un diritto dell'opposizione per tentare di contrastare l'azione della maggioranza e del Governo, a parti rovesciate diventano un risultato dall'esito scontato, al di là della presenza attuale dei senatori in questa seduta. Quindi, credo debbano soccorrere non solo ragioni di natura ordinamentale o regolamentare, ma anche ragione di *fair play*. Il Regolamento prevede che la possibilità di inserimento di un argomento nell'ordine del giorno da parte dell'opposizione abbia lo spazio di una volta ogni due mesi, riservando quindi tutto il resto del tempo al giusto diritto della maggioranza e del Governo di vedere discussi, approvati, respinti o modificati i propri provvedimenti. Ora, nel momento in cui si interviene con una questione sospensiva, che probabilmente avrà successo,

Laseconda considerazione è caratterialmente più legata al provvedimento. Credo che le argomentazioni del senatore Castelli siano state molto significative,

per una apparente democraticità del sistema. L'elezione di giudici, qualunque sia il loro rango e qualunque sia la dimensione delle controversie che essi debbano discutere, introduce un concetto tutt'affatto diverso rispetto all'ordinamento che abbiamo vissuto fino ad oggi nella vita repubblicana e può ventilare ad altri soggetti che non siano giudici professionali reclutati per concorso e con permanenza in carriera fino alla quiescenza in pensione, un potere di giudicare in nome del popolo italiano, traendo da esso stesso, con il suo consenso diretto, tale potere.

che questo dibattito dovrebbe avere. Da questo punto di vista io stesso ho difficoltà ad oppormi in modo netto alla questione sospensiva

della nostra Costituzione, meriterebbe qualche finestra di dibattito televisivo. Infatti, questa sarebbe un'utile occasione per far sapere a tutti i cittadini italiani che la nostra Costituzione anche questa previsione e che loro possono partecipare, se il disegno di legge viene approvato, al processo di formazione dell'ordinamento della giustizia. Sarebbe molto importante per riavvicinare i cittadini al servizio giustizia. Quanto alle considerazioni sul piano del bilancio, si tratta di un'elezione generale diretta, ma la previsione del disegno di legge delega l'ancora all'elezione dei Consigli regionali minimizzandone del tutto i costi, questa elezione avviene nelle stesse sezioni con gli stessi presidenti di seggio e gli stessi scrutatori e prevede una piccola parte di scrutinio aggiuntivo che non comporta un grande onere. Probabilmente è difficilmente quantificabile l'onere in più

un processo culturale che probabilmente spetta a tutti noi accompagnare. Proprio perché sono convinta della proposta e spero che possa passare speditamente, ma anche con un esame approfondito, invito veramente il senatore Castelli ad appoggiare la richiesta di sospensiva.

il primo intervento che si è tenuto in proposito è stato quello del presidente Salvi, il quale ha svolto una sua valutazione in ordine al disegno ed ha espresso un suo parere sulla proposta che ci fosse una più approfondita discussione sul provvedimento. Successivamente all'intervento del presidente Salvi - mi scusi la lunga premessa è intervenuto il senatore Massimo Brutti. Il senatore Massimo Brutti, mi permetterà, rendeva una sorta di dichiarazione spontanea, in quanto riteneva se stesso particolarmente informato sui fatti trattandosi di merito della 2a Commissione. Aggiungeva però, in ordine alle sue considerazioni rispetto al merito della 2a Commissione, alcune considerazioni in ordine alle prerogative della 5a Commissione sullo stesso disegno di legge. In quel caso, il suo essere informato sui fatti aveva una minima *defaillance* precisata dal senatore Albonetti

il collega Brutti non era al corrente che già stamattina era avvenuto un passo in più, come richiesto dal presidente Morando, passo in più che veniva evidenziato dalla proposta che il senatore Castelli avanzava con l'emendamento 1.0.100. La trattazione, quindi, in ordine al parere, reso obbligatorio dal Regolamento del Senato, da parte della Commissione bilancio all'Aula veniva espressa, e quindi superata quella eccezione procedurale. Eccezione che, a questo punto, appariva molto più formale che non sostanziale, atteso che comunque esistono delle formalità che hanno tutta la loro sostanzialità (sembra una formalità che noi si voti in modo ripetuto ogni emendamento con una lungaggine spagnolesca, ma è una sostanzialità evidente perché è il presidio e la difesa della democrazia). Quindi le procedure, *ex* articolo 81, della 5a Commissione rappresentano la difesa che la Commissione fa della Costituzione e quindi il rispetto che quest'Assemblea deve avere nei confronti della Costituzione stessa. Ma cosa succede, Presidente? Che questa formalità ha una sostanzialità molto ristretta in quanto, come osservato in altri interventi, e dal presentatore

può essere benissimo presentato nel corso della discussione dal senatore Castelli in quanto il Regolamento prevede che emendamenti che si rendano necessari per la trattazione del disegno di legge possono essere presentati in Aula, sottoscritti da otto senatori, e che lo stesso parere, ad esempio, visto esempio, visto il contenutissimo rilievo delle risorse occorrenti, potrebbe addirittura essere espresso in Aula, *ex* articolo 100, dal Presidente della Commissione. argomentare in ordine all'articolo 81 e in ordine alle procedure della 5a Commissione ci sembra non un voler riconoscere

faremmo torto al nostro convincimento se non appoggiassimo la richiesta che fa il senatore Castelli di produrci in una votazione contraria alla proposta di rinvio in Commissione.

che programmaticamente non ha alcun intento polemico ma solo l'intento di contribuire a verificare se possiamo, con un rinvio in Commissione come quello proposto dal presidente Salvi, che potrebbe anche essere molto limitato nel tempo, risolvere il problema che a me pare piuttosto complesso e che si pone a proposito - non entro nel merito - della copertura finanziaria del provvedimento. Come il senatore Castelli e gli altri proponenti sanno, il provvedimento, a differenza di quanto affermato

che i proponenti, ben prima che la Commissione bilancio affrontasse il problema, hanno presentato un emendamento che, integrando il disegno di legge (poiché si tratta dei proponenti l'espressione «integrando» non è scorretta), propone una copertura. Se la copertura fosse stata individuata, senatore Castelli, in modo corretto nell'emendamento, avremmo con grande facilità potuto formulare un parere di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'accoglimento dell'emendamento. È però accaduto - lo dico perché la correzione potrebbe essere immediata - che l'emendamento che propone una copertura, quindi riconosce che l'onere c'è e cerca di farvi fronte, è tecnicamente formulato in modo scorretto, perché copre con le disponibilità di bilancio. Lei sa che la legge n. 468 del 1978 non consente di fare una copertura ricorrendo a risorse previste nel bilancio a legislazione vigente, nel presupposto che esse rechino copertura per provvedimenti di legge in vigore e che, intanto, risorse potrebbero essere utilizzate solo in quanto avvenisse una attività di delegificazione che escludesse attività oggi affrontate con le risorse appostate a bilancio. Il risultato, signor Presidente, è che, paradossalmente, se dovessimo immediatamente procedere ci troveremmo in una situazione particolarissima. Abbiamo un disegno di legge su cui complessivamente c'è un parere contrario della Commissione bilancio, bilancio, assolutamente fondato tecnicamente, tanto che gli stessi proponenti hanno affrontato il problema della copertura che nel disegno di legge non è trattato; pertanto su tale disegno di legge c'è un giudizio che determina la sua improcedibilità. Dovremmo quindi paradossalmente provvedere prima ad una votazione che renda procedibile il suddetto disegno di legge, successivamente esaminare emendamenti che affrontino il problema della copertura, ma in questo momento al disegno di legge non è è stato presentato alcun emendamento che rechi la copertura corretta, per cui anche l'emendamento è improcedibile. Secondo me,

riguardo al fatto che, trattandosi di elezione che avverrebbe contestualmente a quella dei Consigli regionali, l'onere è certo ma sicuramente limitato, quindi non mi pare difficile trovare una copertura adeguata, in tempi molto rapidi. Ritengo che i problemi di copertura sarebbero risolti molto facilmente anche attraverso un rinvio in Commissione di pochi giorni che consenta ai proponenti - o ad altri che lo volessero - di integrare la proposta con una copertura corretta, che consentirebbe un parere di nullaosta condizionato. Risolveremmo così il problema della improcedibilità e in questo modo tutto sarebbe più ordinato. Credo che anche i colleghi dell'opposizione che hanno partecipato alla discussione in Commissione bilancio su questo punto

la copertura avanzata sia proponibile o meno. Le posso assicurare però che, dal punto di vista sostanziale, la copertura esiste perché è a valere su fondi previsti sull'ordinamento giudiziario che non è mai entrato in vigore e che sono stati confermati. Basta andare a vedere la Tabella B della finanziaria che voi avete approvato: i fondi ci sono. Vorrei aggiungere, come ultima considerazione, che mi rendo conto, avendolo vissuto più volte, che, non essendo i componenti della Commissione bilancio tutti dei Pico della Mirandola (invece dovrebbero esserlo per la funzione che sono chiamati a svolgere), spesso non riescono a entrare nel merito delle problematiche dei singoli Ministeri: lo dico senza alcuna polemica. Ritorno su un punto che ho già sollevato molte volte: il caso classico è la questione del soprannumero

sullo stesso provvedimento, la nuova Commissione bilancio ha invece dichiarato che era ammissibile a norma dell'articolo 81 della Costituzione. Questo per far capire come, certo non per colpa né del senatore Morando, né degli altri componenti della 5a Commissione, si debbano muovere sulle sabbie mobili, qualche volta

Se si dovesse rinviare, le sedute della Commissione previste per martedì e mercoledì consentirebbero di aprire una finestra già entro mercoledì prossimo. Questo le comunico, tenuto conto certamente della necessità che a decidere sia la Conferenza dei Capigruppo su sua proposta.

che oggi discutiamo, un provvedimento che coinvolge interessi delicati che vanno al di là delle aspettative e degli interessi, di quelli che chiamiamo operatori della giustizia, cioè magistrati, avvocati, personale dell'amministrazione giudiziaria. È un provvedimento che tocca gli aspetti più sensibili dell'azione pubblica, quelli della domanda e dell'offerta di giustizia, e che per questo coinvolge direttamente tutti i cittadini. Ormai da molto tempo alla giustizia si è affidata una parte rilevante delle aspettative di questo Paese: penso agli interventi della giustizia penale che hanno avuto ad oggetto fatti di terrorismo, penso alla dura lotta contro la criminalità organizzata, penso alle indagini e ai processi che hanno individuato gravissime magagne all'interno della pubblica amministrazione. Ma penso anche ai tanti casi in cui ormai si affida al giudice la soluzione di contrasti e dissidi della vita di tutti i giorni (le crisi familiari, la protezione dei minori e dei più deboli, la tutela dei diritti nel mondo del lavoro, del commercio, dei contratti). È interesse di tutti allora - è facile comprenderlo - avere un ordinamento giudiziario che sia a garanzia di una corretta applicazione delle regole e che consenta un'organizzazione funzionale della macchina della giustizia. In questi anni abbiamo avvertito tutti l'esigenza di un cambiamento, di norme più adeguate alle effettive mutazioni della società, ma spesso le risposte sono state condizionate da fattori esterni, da logiche politiche estreme, applicate in una materia che chiedeva solo di essere razionalizzata, adeguata, non orientata a destra o a sinistra. C'è stato uno scontro aspro tra politica e magistratura, che non ha fatto bene al Paese; uno scontro che ha fatto perdere di vista la sostanza,

C'è stato uno scontro aspro tra politica e magistratura, che non ha fatto bene al Paese; uno scontro che ha fatto perdere di vista la sostanza, che ha spinto ad opposti arroccamenti e che praticamente ha messo in crisi il sistema. La risposta deve essere ponderata, meditata, di buonsenso. Va ristabilito il giusto e l'adeguato rispetto per la magistratura nel suo insieme e nei suoi singoli componenti: il rispetto che è dovuto innanzitutto verso chi rappresenta una funzione alta nel nostro ordinamento, quella di interpretare e di applicare le leggi, ma anche rispetto verso chi molte volte ha rappresentato l'ultima frontiera contro l'illegalità e per questo ha pagato anche prezzi altissimi; rispetto verso chi contribuisce con decisioni giuste alla giustizia della vita sociale e privata. Ma accanto a tutto questo non possiamo non rilevare le tante disfunzioni che ci chiedono un intervento deciso: procedimenti lenti, decisioni disomogenee, a volte arbitrarie, disorganizzazione ed inefficienza degli uffici ed inefficienze strutturali. Siamo qui per dare una risposta adeguata, una risposta tesa al miglioramento del sistema; una risposta non contro i giudici né a favore dei giudici, senza pregiudizi, senza tabù, ma soprattutto senza ideologismi. Stiamo discutendo e stiamo per votare un testo che rappresenta una risposta seria e di buonsenso a un problema che abbiamo definito strutturale. Il testo proposto dal Governo e parzialmente modificato dalla Commissione giustizia è frutto di un lavoro intenso e faticoso, di una discussione e di un confronto serrato tra i diversi orientamenti, una soluzione forse non perfetta - alcuni aggiustamenti sono ancora necessari - ma un grosso passo avanti nello spirito corretto della ricerca di strumenti di miglioramento. Credo che un primo punto da sottolineare sia lo sforzo di accrescere la competenza e la professionalità dei magistrati, a partire dalle regole per l'accesso in magistratura.

ha garantito fino ad oggi che i magistrati fossero scelti tra i giovani, non solo quelli più capaci e competenti, ma anche i più motivati proprio perché la durezza della prova imponeva un percorso di studi lungo e praticamente esclusivo. però tutti constatato che di anno in anno il concorso si è fatto sempre più affollato, tanto che si sono dovuti studiare meccanismi di preselezione, i *quiz*, che però non garantivano, né l'equità, né l'efficacia del risultato di scrematura. Con questo provvedimento si dà una risposta decisamente più seria, imponendo che i candidati al concorso, che naturalmente resta completo e impegnativo (anzi, un po' più impegnativo, con l'inserimento della materia del del diritto fallimentare e del *test* di lingua straniera), debbano aver compiuto, dopo la laurea, un'esperienza professionale di approfondimento degli studi molto significativa. Un concorso che diviene di secondo grado e che garantisce che possano accedervi giovani che abbiano già una formazione, senza che le domande e le prove di chi non é motivato, né preparato appesantiscano le procedure di valutazione. D'altra parte, mi sembra che l'ampia gamma di esperienze pregresse richieste consenta di accedere al concorso sia a chi dopo la laurea preferisce concentrarsi sugli studi, frequentando scuole di specializzazione o dedicandosi alla ricerca universitaria, a chi preferisce o deve svolgere un'attività lavorativa, come ad esempio nella pubblica amministrazione o nella libera professione forense, o comunque retribuita, come quella del magistrato onorario (colgo qui l'occasione per apprezzare la considerazione che si è dedicata a questa importante funzione, che va opportunamente valorizzata, accanto al ruolo della magistratura togata). Sulla stessa linea di quanto appena detto, volevo sottolineare l'importanza della norma che prevede che nel primo periodo di esercizio delle funzioni non si possano svolgere più quelle funzioni delicate o di maggiore impatto che comunque richiedono un'esperienza consolidata, come ad esempio quelle del GIP, del GUP e del giudice penale monocratico. Credo sia un segnale forte l'aver inserito in tale norma le funzioni requirenti; una giustizia più giusta passa anche da qui, dall'affidare l'attività requirente e investigativa a magistrati non solo teoricamente preparati, ma anche capaci e adeguatamente formati. Non bastavano, e ne eravamo consapevoli tutti, i pochi mesi di tirocinio a garantire quella competenza, quella ponderazione e quella capacità che l'attività del pubblico ministero richiede, soprattutto nelle zone più difficili del Paese o per reati particolari per i quali il momento delle indagini è importantissimo e delicatissimo. Ancora, è da salutare con favore la rigorosa disciplina che riguarda la valutazione della professionalità dei magistrati. È una disciplina che era divenuta urgente e ormai improrogabile. All'attribuzione di funzioni sempre più delicate deve corrispondere una professionalità alta e diffusa, in tutti i gradi e le sedi giudiziarie. È un giudizio condiviso anche dalla magistratura associata, che verifica ogni giorno come alcuni, forse pochi, magistrati improduttivi, inadeguati e svogliati hanno spesso fatto pagare un prezzo alto in termini di credibilità ai magistrati che lavorano invece con dedizione e capacità. È un'esigenza che tutti sentiamo impellente, operatori della giustizia e cittadini comuni, che non poteva trovare una risposta troppo rigida, che mortificasse l'attività quotidiana dei giudici, che li costringesse ad esami, concorsi e valutazioni, magari distogliendoli dal lavoro ordinario, prezioso per tutti gli utenti. Appare equa, a mio parere, la proposta contenuta nel testo che stiamo discutendo e che prevede una valutazione completa fatta secondo parametri ben precisi, elencati analiticamente secondo profili che individuano gli aspetti essenziali dell'attività del magistrato e cioè la capacità professionale, la laboriosità, la diligenza, l'attitudine alla dirigenza; capacità questa che non deve più ritenersi automaticamente acquisita dopo un certo numero di anni di attività, ma che deve essere appositamente dimostrata. Va apprezzata anche la disciplina che interviene sul tema della temporaneità delle funzioni; anche questo è un aspetto dove la riforma appariva urgente sia per evitare incrostazioni di potere da parte di magistrati che per un periodo lunghissimo ricoprono certi incarichi, soprattutto se delicati ed esposti penso ai giudici fallimentari, ad esempio - sia per evitare forme di pigrizia professionale, di *routine* che a lungo possono prevalere su un'attività seria e attenta alle evoluzioni della società e del diritto. Apprezzo soprattutto il principio della temporaneità delle funzioni direttive che è stato definito secondo modalità che non ledono i legittimi interessi dei magistrati a ricoprire posti dirigenziali e a fare carriera, né pregiudicano l'interesse a che la permanenza a capo di un ufficio non sia troppo breve così da impedire di far tesoro di un'esperienza maturata, ma salvaguarda l'esigenza di un corretto ricambio nelle posizioni di vertice, dove più facilmente possono annidarsi situazioni di potere. Questa riforma, questo provvedimento, dopo mesi di critiche, scontri e polemiche, seguiti da un periodo di ascolto e rispetto reciproco tra politica e magistratura, rappresenta l'occasione per sancire un metodo, la ripresa di una collaborazione che dovrebbe essere intensa e proficua nell'interesse del Paese intero.

sono dedicate ai criteri fondamentali da perseguire nell'impegno di intervenire con provvedimenti di riordino dell'ordinamento giudiziario ispirati al rispetto degli equilibri costituzionali e dell'indipendenza della magistratura come strumento di tutela dei diritti dei cittadini. Un primo passo è stato compiuto lo scorso autunno ed ora spetta alle Camere, ed anzitutto alla maggioranza, di dare piena attuazione a quell'impegno entro il 31 luglio. La posizione di indipendenza che la Costituzione riconosce ad ogni soggetto che eserciti funzioni giurisdizionali non esclude che il giudice si presenti in ogni caso come «soggetto alla legge», in ossequio al basilare principio di legalità. L'indipendenza del giudice, che la riforma dell'ordinamento assicura attraverso le norme funzionali ed organizzative, non significa arbitrio, bensì libertà di interpretazione dei testi normativi, nell'ambito però di un sistema precostituito. Proprio attraverso la soggezione alla legge, che il giudice attua in piena autonomia organizzativa e in totale indipendenza funzionale, il magistrato può cogliere l'essenza delle tensioni sociali espresse dalla legge medesima. Dare un assetto funzionale ed efficace alla magistratura consente quindi di evitare la tentazione di facili scorciatoie come quelle che oggi, di fronte ad una percezione di insicurezza da parte dei cittadini, fanno risuonare sempre più forti gli inviti alla legislazione d'emergenza, all'inasprimento delle pene, alla cancellazione dei benefici carcerari o, nei casi peggiori, alla svolta repressiva dei fenomeni e dei conflitti sociali che abbiamo di fronte. Il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario presentato dal ministro Mastella, come modificato dalla Commissione giustizia, certamente non esaurisce tutte le problematiche oggetto di discussione in questi ultimi anni ed è quindi suscettibile di miglioramenti in sede parlamentare, ma crediamo sia indispensabile giungere ad approvare in tempo utile un testo che, avvalendosi anche di un contributo non ostruzionistico dell'opposizione - questo almeno è stato in Commissione e nella sottocommissione il pregio di affrontare i nodi fondamentali attorno ai quali costruire, con i successivi decreti delegati, un percorso di ricostruzione dell'ordinamento. Si tratta, in particolare, della riforma del concorso d'accesso alla magistratura, del rapporto tra il magistrato di nuova nomina con le funzioni di pm o di gip, del delicato equilibrio delle funzioni fra magistratura giudicante e magistratura inquirente, con adeguati bilanciamenti nel caso di passaggio da una funzione all'altra, del passaggio dai rischi di un sistema imperniato sul concorsificio per l'avanzamento di carriera all'introduzione di criteri adeguati per una necessaria valutazione periodica della professionalità, nonché della salvaguardia delle valutazioni proprie del CSM sulla carriera dei magistrati e della previsione della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi. Il lavoro svolto in Commissione, pur faticoso, ha portato ad un testo equilibrato che offre alle Camere, e quindi al Governo come organo delegato, criteri e princìpi fondamentali da attuare tempestivamente per dare concretezza ai princìpi di autonomia e indipendenza della magistratura che la Costituzione riconosce a tutela del servizio pubblico della giurisdizione da rendere ai cittadini. I tempi della giustizia costituiscono oggi un fattore cruciale per dare corpo al bene comune rappresentato dall'amministrazione della giurisdizione. La necessità di una rapida approvazione della riforma va quindi accompagnata ad un intervento per riequilibrare lo stato critico delle dotazioni degli uffici giudiziari ed affrontare il problema delle risorse e dei mezzi. Il contributo che questa riforma può offrire consiste nel delineare un sistema fondato su una consapevole e responsabile salvaguardia, sul piano sostanziale e sul piano formale, dei fondamentali valori di autonomia e di indipendenza dell'ordine giudiziario in cui la formazione dei magistrati dovrà essere centrale e le scelte dei candidati che andranno a ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi saranno frutto di accertate professionalità e di sperimentate qualità. Spetta infatti ai dirigenti degli uffici (requirenti e giudicanti) l'adozione di iniziative e provvedimenti idonei a razionalizzare la trattazione degli affari, nel rispetto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e di quello della soggezione di ogni magistrato esclusivamente alla legge, ma anche dei principi consacrati dall'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento della pubblica amministrazione. A questo proposito, una più incisiva diffusione di una comune cultura organizzativa poggia inevitabilmente sulla necessità di evitare il vuoto e la conflittualità che possono sorgere da una mancata approvazione della proposta all'esame del Parlamento, come ha recentemente rilevato davanti al CSM lo stesso Presidente della Repubblica. Lo stralcio di alcune parti del provvedimento operato dalla Commissione ha consentito di concentrare l'attenzione su una serie di priorità per rafforzare gli organi ai quali è affidata l'amministrazione della giustizia nella materia civile e penale, lo stato giuridico dei magistrati che esercitano la giurisdizione ordinaria e che nel loro complesso costituiscono l'ordine giudiziario, e la composizione e struttura degli organi e degli uffici giudiziari. In questa sede sono previste articolazioni e stabilite le funzioni, oltre che la condizione giuridica soggettiva dei magistrati, comprensiva della carriera, dei diritti e delle guarentigie di indipendenza, dei doveri e delle responsabilità. Non dimentichiamo che l'ordinamento, secondo una consolidata giurisprudenza sia della Corte costituzionale che della Cassazione, si inserisce in un più ampio contesto nel quale è oggi vigente un complesso di atti normativi che hanno un carattere ben diverso da quello di norme di mera interpretazione della disciplina legislativa; si pensi, in particolare, all'attività del CSM le cui deliberazioni, circolari, istruzioni investono tutti i settori dell'ordinamento giudiziario e costituiscono ormai un *corpus* normativo di notevolissima portata e di indiscutibile rilevanza. Pertanto, si comprende come non sia più differibile, da parte della politica, la rinuncia ad aggiornare l'ordinamento, assicurando l'attuazione dei principi fondamentali: il riconoscimento del potere giudiziario come autonomo ed indipendente da ogni altro, l'esclusione di ogni gerarchia di tipo burocratico fra i giudici, l'esclusione di ogni dipendenza nei confronti di qualunque autorità che non sia quella della legge. L'esercizio dell'attività giurisdizionale attualmente diffuso fra una pluralità di giudici i quali sono reciprocamente indipendenti. Il problema di conciliare l'esigenza di salvaguardare il carattere diffuso della funzione giurisdizionale con quella di assicurare l'autonomia e l'indipendenza del potere giudiziario da ogni altro potere ha trovato una soluzione efficace nell'assegnazione ad un organo non giurisdizionale ma nettamente separato dal potere esecutivo della generalità delle funzioni capaci di influire sullo *status* del giudice e del pubblico ministero, strumentali rispetto all'esercizio della giurisdizione, funzioni che prima dell'avvento della Costituzione erano attribuite al Ministro Guardasigilli cui attualmente è invece riservata la titolarità dell'azione disciplinare, sia pure in via non esclusiva, e con essa il compito di assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Il disegno di legge delega riesce a trovare su questo punto, anche a seguito delle modifiche intervenute in Commissione, un equilibrio soddisfacente proprio con riferimento alla struttura pluralistica e ai compiti del CSM, dal momento che il noto principio della divisione dei poteri non può determinare una contrapposizione tra i poteri stessi e ciò è possibile con un buon funzionamento del sistema di autodisciplina interna, realizzato attraverso i meccanismi di autogoverno che deve contemporaneamente assicurare l'indipendenza interna dei magistrati, non solo rispetto al potere esecutivo. Positive sono le soluzioni individuate per la selezione e la formazione professionale dei magistrati, in modo da rafforzare una cultura professionale tendenzialmente omogenea fondata sulla valutazione dell'idoneità e dell'attitudine e in collegamento con i Consigli giudiziari, allo scopo di incentivare il dialogo con la classe forense e nella convinzione che i valori costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza del giudice non debbano comportare forme di isolamento della magistratura, senza cadere negli equivoci della composizione mista. Su questi aspetti, come anche sui profili essenziali del reclutamento e del procedimento disciplinare, connesso strettamente alle garanzie di indipendenza interna, occorre che ogni schieramento politico offra un proprio contributo: questo è stato l'orientamento della Commissione giustizia, per cui è essenziale che l'articolato lavoro espresso in quella sede non sia vanificato da un atteggiamento meramente ostruzionistico o aprioristicamente contrario, alla luce dell'interesse del Paese ad avere un ordinamento giudiziario forte, nell'ottica di bilanciamento tra poteri. La Commissione ha ascoltato le voci della magistratura organizzata, così come dell'avvocatura, in materia di separazione delle funzioni. Le soluzioni individuate sono ovviamente migliorabili, ma sempre nella consapevolezza che per avere un ordinamento giudiziario forte ed indipendente è necessario dotare la Repubblica di un *corpus* aggiornato di regole e norme capace di rafforzare gli aspetti costituzionalmente rilevanti dell'imparzialità e professionalità dei magistrati cui è connesso il principio di precostituzione del giudice, ed è bene che tale opera sia svolta dalle Camere in tempi tali da non rendere necessario il ricorso alla decretazione d'urgenza.

il disegno di legge, nel testo approvato dalla Commissione, che viene oggi al nostro esame, rappresenta certo un miglioramento rispetto all'originario disegno di legge governativo; non possiamo, inoltre, non sottolineare positivamente il fatto che rispetto ai *diktat* dell'Associazione nazionale magistrati,

Di questo diamo realmente atto in particolare al relatore, senatore Di Lello. Ma questo non ci induce a un giudizio positivo sul testo che stiamo discutendo non tanto e non solo perché vi sono alcune norme che destano motivi di perplessità, ma per una più generale considerazione sulla forma e sui modi con cui si è affrontato e si affronta il problema dell'ordinamento giudiziario e quello più in generale della collocazione della magistratura nel nostro quadro costituzionale. Mi soffermerò innanzitutto su una questione che più direttamente inerisce al provvedimento al nostro esame. L'attuale testo prevede la possibilità di passare dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa per ben quattro volte nel corso della carriera. Si tratta, evidentemente, di una soluzione che pregiudica la possibilità di distinguere il ruolo e la funzione del pubblico ministero da quella del giudice, come invece esigerebbe il dettato costituzionale che, all'articolo 111, esplicitamente prevede che il giudice sia terzo e imparziale. Consentire il tramutamento delle funzioni per ben quattro volte nel corso della carriera di un magistrato equivale ad annacquare il timido barlume di separazione di funzioni, posto che già oggi, mediamente, un magistrato passa da una funzione all'altra due o tre volte nell'arco della propria carriera. Se questa previsione legislativa non è accettabile (e in merito ho presentato con i colleghi Biondi e Ziccone delle proposte emendative), va invece apprezzata la norma che stabilisce che non solo i giudici che non hanno funzioni direttive o i sostituti del pubblico ministero debbano cambiare distretto al momento del passaggio di funzione (come faceva l'originario testo governativo), ma che tale obbligo sia esteso a tutti i magistrati (anche a coloro che ricoprono funzioni direttive) e che i magistrati che lavorano nelle cinque Regioni che hanno più di un distretto di Corte d'appello debbano uscire dalla Regione per cambiare funzione. Ma al di là di questo aspetto, come dicevo, si pone la questione di una più generale riflessione su come debba essere risolto il problema di un migliore funzionamento del nostro sistema giudiziario. Ho già avuto occasione di affermare, nel corso del dibattito sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, presentata nella scorsa legislatura dall'allora ministro Castelli, che il nostro sistema giustizia è caratterizzato da due diversi mali: da un lato, la condizione di conflittualità dell'ordine giudiziario con gli altri poteri dello Stato, dall'altro, una ormai congenita inefficienza, specie nel settore del contenzioso civile. E come pertanto vi sia bisogno, non solo di un intervento del legislatore ordinario, ma anche di una revisione costituzionale. Sul primo punto, relativo alla separatezza, confinante con l'ostilità, che la magistratura associata ha assunto rispetto al potere politico, se separatezza volesse dire anche orgogliosa rivendicazione della propria autonomia (e in particolare dell'autonomia del singolo giudice) *nulla quaestio*. Ma se la separatezza confina con l'ostilità, in nome di un presunto primato morale, questo esce dal quadro costituzionale. Qui si pone il delicato problema dell'autogoverno della magistratura e della revisione costituzionale delle norme, che questo disegno di legge ordinario non può toccare, sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura. È un tema che fu già oggetto di scontro già alla Costituente, in contraddittorio con la tesi dell'onorevole Scalfaro, che poi prevalse, l'onorevole Togliatti e l'onorevole Laconi sostennero che il Consiglio superiore della magistratura avrebbe dovuto essere "un organismo il quale assume una funzione particolare di antidoto alla completa autonomia del potere giudiziario come tale", il che li portava a ritenere che il Consiglio superiore dovesse formato per metà da magistrati e per metà da membri eletti dall'assemblea nazionale: un elemento - secondo Togliatti - che accresceva, non diminuiva, il prestigio della magistratura. Dicendo questo, non voglio sposare la tesi che in allora sosteneva la sinistra, ma credo si debba riflettere, per superare la separatezza, sull'ipotesi di un Consiglio superiore della magistratura modellato su uno schema analogo alla Corte costituzionale, da tempo ipotizzato dal collega Maccanico, vale a dire di un terzo di nomina dei magistrati, un terzo del Parlamento ed un terzo del Capo dello Stato, anche nel suo ruolo di Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Il secondo punto che ho sottolineato è relativo relativo alla necessità di realizzare un recupero di efficienza che garantisca ai cittadini la tutela dei propri diritti in tempi e con metodi accettabili. La soluzione ordinamentale che appare più logica è la responsabilizzazione dei vertici degli uffici. dei vertici degli uffici. Si tratta di dare ad essi reali poteri dì direzione e di controllo. In questo senso, penso occorra introdurre un secondo comma all'articolo 97 della Costituzione, prevedendo che il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, i presidenti e i procuratori generali presso le corti d'appello, i presidenti e i procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari assicurino, ciascuno nel proprio ambito di competenza, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia secondo i criteri di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Inoltre, ed è una provocazione che lancio e che si ricollega in qualche modo al dibattito che abbiamo avuto poc'anzi, bisognerebbe forse anche riflettere sull'ipotesi di soluzioni diverse tramite l'elezione popolare per le designazioni dei responsabili delle corti d'appello, dei tribunali e delle procure; che poi non è tanto una novità se, come ricorda Carlo Lozzi nel saggio «La magistratura innanzi al nuovo Parlamento» del lontano 1883, già il procuratore Giuseppe Manfredi, che poi fu presidente di questo ramo del Parlamento, nel discorso avanti alla Corte di cassazione di Firenze - allora vi era la pluralità Corti di cassazione - aveva sostenuto «il radicale innovamento della elezione popolare dei giudici", opinando che "il sistema da propugnarsi debba essere tale da conciliare il principio dell'elezione con quello dell'autonomia propria dell'ordine giudiziario!». Colleghi senatori, le brevi considerazioni che ho voluto esporre sono solo alcune sollecitazioni per una più approfondita riflessione sui problemi complessi del nostro ordinamento giudiziario

da poco faccio parte di questo altissimo consesso e devo dire che ho avuto esperienze più negative che positive. L'esperienza veramente positiva, la prima,

Credo che mai all'interno della nostra Commissione si sia lavorato con tanta serenità, con tanto impegno e con tanta competenza. Ognuno di noi, sia della maggioranza che dell'opposizione, ha cercato di dare il meglio di se stesso, il meglio della propria professionalità,

ciascuno di noi aveva compreso ed aveva piena consapevolezza che l'ordinamento giudiziario non è fatto e non poteva essere fatto né nell'interesse degli avvocati, né nell'interesse della magistratura; l'ordinamento giudiziario è un complesso di norme che viene fatto soprattutto nell'interesse della giustizia - con la lettera maiuscola

la cui giunta si è dimessa, e che forse proclamerà uno sciopero, ed ha lasciato insoddisfatti anche gli avvocati. Nella mia vita di magistrato ricordo di essere stato qualificato politicamente nei modi più diversi ed opposti.

Abbiamo conseguito risultati ottimi, sui quali ci siamo trovati tutti d'accordo. Innanzitutto, nonostante questo sia ancora oggi il motivo dello sciopero degli avvocati, abbiamo uniformemente rigettato la separazione delle carriere. Persino la legge Castelli aveva rifiutato tale separazione ed io credo che noi l'abbiamo rifiutata per una ragione molto semplice:

Quindi, separazione delle carriere per coloro che la sostengono significa, soprattutto, sottoposizione del pubblico ministero all'Esecutivo. Sotto questo profilo abbiamo avuto un'esperienza estremamente negativa durante il Ventennio e quindi, non a caso, l'abbiamo abbandonata. abbandonata. Tale esperienza negativa purtroppo ha avuto ripercussioni anche dopo, perché nonostante sia intervenuta la nostra Costituzione a stabilire l'indipendenza della magistratura, sia come magistratura giudicante che requirente,

della sottoposizione del pubblico ministero all'Esecutivo sono stati notevoli. Credo vada ricordato, a proposito di questa sottoposizione, un istituto che ha scosso fortemente l'opinione pubblica quando è stato impiegato, cioè la rimessione per legittima suspicione. la rimessione per legittima suspicione. Essa fu, in questa Repubblica, adottata per la prima volta in occasione di una tragedia terribile, quella del Vajont, in cui morirono ben 2.000 persone e il processo fu trasferito dal procuratore generale di Venezia a L'Aquila, con le conseguenze che tutti noi sappiamo:

rimessione per legittima suspicione, ho avuto occasione di vedere una circolare del lontano 1939 in cui il Ministro fascista si lamentava con i procuratori generali perché facevano eccessivo ricorso a questo istituto. istituto. La circolare, in cui si diceva che era disdicevole fare ricorso a tale istituto perché poteva indurre le persone a ritenere che la magistratura fosse sottoposta all'Esecutivo e, sopratutto, ancora più disdicevole perché poteva far ritenere che si potesse ottenere sentenza diversa cambiando i giudici, i giudici, era l'indice sicuro di quanto la magistratura requirente avesse subito l'influenza non solo dell'Esecutivo, ma anche del mondo politico periferico, dei gerarchi periferici, tanto da essere indotti a richiedere la rimessione per legittima suspicione e a farne persino abuso per casi che tale rimessione non richiedevano.

devo dire che questa Assemblea deve tener conto del fatto che la proposta avanzata dal Ministro di consentire anche ai laureati con un'alta votazione con un'alta votazione di accedere immediatamente alla magistratura non è stata accolta dalla Commissione, perché si è ritenuto che il voto di laurea, per le differenze esistenti tra le varie università nel valutare gli allievi, potesse essere non decisivo dell'ottima qualità del laureato quindi si potessero creare disparità di trattamento tra laureati in una università e in altre, molto più larghe Pertanto, a questo punto, forse sarà il caso, al più presto possibile, di prendere in seria considerazione la riforma universitaria.

non attribuire le funzioni monocratiche, che sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice unico di primo grado, oltre che quelle di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, a coloro che non avessero superato la prima valutazione, che avviene dopo quattro anni. Questa, secondo me, è stata una grande conquista e dimostra quanto affermavo all'inizio, e cioè che noi abbiamo operato in Commissione soprattutto nell'interesse della giustizia e dei cittadini. Abbiamo operato non tenendo in alcuna considerazione i privilegi di corporazione e quindi per la prima volta si potrà evitare che soprattutto nelle sedi disagiate possano andare allo sbaraglio magistrati di prima nomina,

che i magistrati non possono restare nelle sedi disagiate che, come sapete, vengono stabilite dal Consiglio superiore della magistratura,

di sedi disagiate facciano domanda di trasferimento, vengano privilegiati nel trasferimento dinanzi a tutti coloro che si trovano a fare domanda per la stessa sede. In questo modo abbiamo ottenuto il risultato di incentivare i magistrati che hanno già superato la prima valutazione ad andare nelle sedi disagiate

importante e decisiva è stata quella della temporaneità delle funzioni direttive che avevamo auspicato da tanto tempo e che finalmente è stata attuata, a mio avviso nella maniera migliore. non solo è stato stabilito che le funzioni direttive, che durano quattro anni, possono essere rinnovate una sola volta, ma è stato altresì deciso che, quando scade il primo quadriennio, per il titolare dell'ufficio direttivo entri in concorso con gli altri magistrati e che quindi competa, anche se poi, nell'ipotesi di parità in graduatoria, sarà privilegiato rispetto all'altro. Il senatore Castelli accennava al trattamento diverso che ci sarebbe stato per la conferma di chi non viene nominato nella stessa sede anche in soprannumero.

trovarsi in una condizione di disagio economico per questo. Molto probabilmente il posto vacante ci sarà sempre e, se non ci sarà in quel momento, sarà facilmente raggiungibile e comunque non ci sarà una questione economica,

potrà esercitarla anche in soprannumero, per l'arretrato che tutti quanti sanno esserci presso i nostri uffici giudiziari. Altra misura che è stata adottata è il miglioramento della pur congrua ed articolata disciplina che era stata stabilita dal Ministro per quanto riguarda la valutazione dei magistrati ai fini della progressione nelle funzioni. Anche in questo caso il miglioramento è stato fatto introducendo introducendo criteri oggettivi che devono essere indicati specificamente dal Consiglio superiore della magistratura, in modo da creare una uniformità di valutazione da parte di tutti i Consigli giudiziari

critica che è stata ripetuta ancora oggi dal collega Del Pennino, è di aver dato la possibilità di quattro variazioni:

il primo periodo non sarà valutato in questo cambio di funzioni. Soprattutto bisogna tener conto che tale previsione non incide in maniera estremamente negativa sulla necessità di doversi spostare da un distretto

giudicante. Pertanto, se qualcuno ha delle esigenze di rimanere in una sede, può sempre restare o nella funzione requirente in cui già è, o in quella giudicante in cui già si trova, aspettando poi un'occasione migliore per far

ed è per questo che invito il senatore Di Lello a fare ricorso alla sua pazienza, almeno per il tempo del mio intervento,

Secondo ragioni di cortesia, assicuro fin d'ora il senatore Di Lello che non abuserò della sua pazienza. Proclama: «Io sto con i magistrati che lavorano e non con quelli che impediscono loro di lavorare o li criminalizzano». È un proclama del ministro Di Pietro, il quale ha altresì ritenuto di affermare che in Commissione giustizia si era realizzato un inciucio, cioè qualcosa che, pur scontando il suo pittoresco linguaggio, non può essere assimilato a quell'invito al confronto che pure era stato mosso dal Capo dello Stato. Un inciucio: ci spiegasse il ministro Di Pietro che cosa noi del centro-destra abbiamo dato al centro-sinistra e che cosa il centro-sinistra ha dato a noi del centro-destra. Più in particolare, ci spiegasse quale cointeressenza tra centro-destra e centro-sinistra vi sia stata per arrivare al testo varato dalla Commissione. La realtà è che spesso taluno fa dei ragionamenti dietrologici, o meglio, taluno, attraverso la dietrologia, cerca la strada della suggestione e della propaganda, quasi che, in questo Paese, il livello medio dell'intelligenza fosse particolarmente basso e il popolo italiano non fosse ormai avvertito di questi giochi tipicamente politici che tanto allontanano la cittadinanza dalla politica. politica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vedete, se dovessi ragionare secondo la dietrologia che mi pare permeare i recenti interventi del ministro Di Pietro, direi subito che, che, a fronte di acquisizioni molto antiche, mi sembra particolarmente strana la coincidenza temporale in base alla quale ieri il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato, sia pure all'unanimità, un testo che affronta una questione risolvendola in punto di fatto, senza un'acquisizione completa e senza sentire le varie parti in causa: secondo questa

con buona pace del senatore D'Ambrosio, al quale do atto della correttezza del suo intervento circa gli eventuali miglioramenti che in Aula si potrebbero apportare

Uno sciopero, quello dell'Associazione nazionale magistrati, che, a sentire le parole del consigliere Rossi, esponente di punta della magistratura associata, sembrerebbe incentrarsi su due punti: primo, la cosiddetta separazione delle funzioni; secondo, le norme, oggetto di un proposta di stralcio, che tendono a un ritorno indietro, con riferimento alla struttura dell'ufficio del pubblico ministero.

perché scontenta sia l'Associazione nazionale magistrati, sia gli avvocati. Lo sa, senatore D'Ambrosio, che la stessa identica cosa dicevamo noi quando abbiamo varato la riforma Castelli? È un ottimo testo, perché scontentando l'Associazione nazionale magistrati e gli avvocati, non ha preso le parti né dell'una, né dell'altra, ma ha tentato la ricostruzione di un sistema, la più neutrale possibile. E allora, trovandoci nella stessa, identica situazione, mi chiedo quale dei due testi, il vostro o il nostro, sia migliore. Certo, di quella tanto vituperata riforma Castelli, che tanti scioperi - ahimè - ha subito o, meglio, ha stimolato nell'ambito dell'Associazione nazionale magistrati, gran parte è già in vigore.

quegli scioperi finalizzati proprio a non far entrare in vigore anche quella parte che con il vostro accordo è entrata in vigore. Noi non siamo soddisfatti del testo varato dalla Commissione, pur riconoscendo che qualche punto, sia pure in termini minimali, soddisfa talune nostre esigenze, o meglio, soddisfa talune esigenze del Paese. Certo è però che - così - così lo diciamo in chiaro nell'ambito dei lavori parlamentari, affrontando il primo dei problemi che conseguirà da questa vostra riforma voi costruite il concorso in magistratura come un concorso di secondo grado, cioè sostanzialmente come un concorso similare al concorso per la giustizia amministrativa e per la magistratura contabile. Ma questo vi pone il primo problema, fondamentale, enorme: adeguerete o no le retribuzioni e le progressioni in carriera della magistratura ordinaria a ciò che è attualmente previsto per la magistratura amministrativa e contabile? È evidente È evidente che se ciò non farete - e credo non lo potrete fare per un problema di copertura finanziaria - creerete una inaccettabile disparità di trattamento all'interno delle magistrature, che hanno un'analoga modalità di entrata: il concorso di secondo grado. Non solo, ma con il successivo effetto di veicolare verso la magistratura amministrativa e contabile, per evidenti ragioni sia economiche sia di carriera, se così si può dire, le menti migliori i nostri giovani laureati in giurisprudenza. Davvero non vi sarebbe senso per un giovane particolarmente preparato, salvo vocazioni innate, di accedere ad una carriera sotto il profilo economico e sotto il profilo della progressione più mortificante rispetto ad analoghe carriere. Il problema c'è, e lo dovrete affrontare proprio con la categoria dei magistrati che per molto tempo sono stati mortificati. Sono stati mortificati, ad esempio, quando in magistrature similari si è consentito, come tuttora si fa, di arrivare da giudice di tribunale al secondo livello a presidente di sezione di Cassazione parlo della questione economica - in soli dodici anni quando per i magistrati ordinari ne abbisognano ben ventitré ancora. Ma questo è un vostro problema! Certo è che quando si costruisce un sistema, esso non rimane avulso dall'intero ordinamento; provoca delle conseguenze anche sui settori vicini. E questa è la prima conseguenza con cui voi vi dovrete misurare. Distinzione delle funzioni: credo che quello che avete scritto nel testo varato dalla Commissione sia quanto di più si poteva ottenere sulla pressione della magistratura associata e su un certo appiattimento registrato da parte del Ministero della giustizia sulle posizioni della magistratura associata, in termini di distinzione delle funzioni. Non a caso, l'Associazione nazionale magistrati lamenta esattamente queste distinzioni. Trovo davvero una ipocrisia davvero una ipocrisia questa storia del numero delle volte per le quali è consentito il passaggio da una funzione all'altra.

cambiando sempre distretto. Capite da soli che questo appartiene alle ipotesi del terzo tipo, cioè non avverrà mai, così come non avviene attualmente. Fate una norma di facciata, e l'Associazione nazionale magistrati, che ben conosce il sistema, darà delle dimissioni di facciata.

sicuramente coartati, il primo in ragione del posto in graduatoria, il secondo teso ad un riavvicinamento alla sede di provenienza.

per tutta la sua carriera ha fatto il giudice, essendo stato solo per cinque anni procuratore della Repubblica e, viceversa, per l'incarico di presidente di tribunale. Il che, evidentemente, essendo libero l'accesso agli incarichi direttivi requirenti e giudicanti, svuota di contenuto oggettivo la vostra inimmaginata separazione delle funzioni. Certo, è meglio di niente, ma la separazione delle funzioni, ha ragione il senatore D'Ambrosio, che avevamo in modo diverso, se mi consente, più chiaro, forse più *tranchant,* inserito anche nella riforma Castelli, è una richiesta che oggettivamente viene dal popolo italiano; e di questo i magistrati si devono rendere conto. Non è più possibile per la gente vedere chi ieri sosteneva l'accusa dal banco del pubblico ministero sedersi il giorno dopo nella stessa aula nel banco del giudice. Non è più possibile: e di questo i magistrati si devono rendere conto, perché la realtà è che se i magistrati continuano a fare quadrato sui loro privilegi e sulle loro rendite di posizione, produrranno un danno enorme alla magistratura nel suo complesso, a una magistratura che, diciamocelo una volta per tutte, per oltre il suo 90 per cento, è costituita da professionisti di assoluta onestà, trasparenza e capacità, e che per troppo tempo è andata alla deriva per colpa di pochi,

anomali di magistrati, che spesso sono stati oggetti della protesta dei magistrati stessi? Ricorda quando si parlava della registrazione dell'interrogatorio del detenuto in carcere?

Le cose sono andate avanti; l'unico inconveniente fu che tre o quattro mesi dopo, in quel di Tortona, si scoprì che un interrogatorio verbalizzato era completamente difforme dalla registrazione; non solo, ma si scoprì che, proprio per evitare tale difformità, qualcuno aveva immaginato di operare delle manipolazioni sulle bobine. Quando si fa una riforma, non la si fa per un capriccio personale; la si fa perché le cose così come sono non vanno bene, e attraverso la riforma si cerca di modificare un sistema, non per danneggiare Tizio o Caio, ma per rendere quel sistema sicuramente più funzionale. Questo dovrebbe essere lo scopo della riforma, e confesso che, sotto il profilo della separazione delle funzioni, sia pure in termini minimali, il testo varato dalla Commissione coglie nel segno e spero, con l'accoglimento di taluni emendamenti, che possa cogliere ancora più nel segno.

che quel giudice non ha relazioni di corridoio con altri uffici e che, quindi, la sua decisione attraverso il rito, che non a caso si celebra con la toga, potrà essere accettata. Ma per il resto in che cosa voi modernizzate il sistema? Ho detto che non voglio abusare della pazienza del senatore Di Lello Finuoli, onde per cui cerco di andare rapidamente alla conclusione. progressione in carriera, ma qual è la novità? Che ogni quattro anni valuterete i magistrati? E con quali strumenti nuovi li valuterete? Ma andate a vedere le relazioni che riguardano i magistrati: sono tutti Carnelutti, tutti Calamandrei. Ma è possibile che non vi sia un rapporto, una relazione nei confronti di un magistrato che affermi che questo magistrato, tutto sommato sì, il diritto lo conosce, ma non ne ha una conoscenza eccezionale? E perché sono tutte così? Diciamocelo fino in fondo: perché solo l'omogeneità delle relazioni consente un esercizio smodato del potere discrezionale valutativo da parte del Consiglio superiore della magistratura. E poi gli incarichi che sono ad esse correlati: veramente vogliamo discutere di come vengono dati gli incarichi dal Consiglio superiore della magistratura? Davvero vogliamo dirci le reali ragioni per cui un determinato posto attende per un anno, due anni, la nomina dell'incarico direttivo, e quella nomina avviene quando si liberano posti similari, quindi tutti i giochi di corrente sono pronti? Voi, con questo sistema, non toccate - lo sottolineo,

non garantite l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati al loro interno, che è quella che i magistrati sentono molto di più, perché, vedete, noi magistrati non siamo particolarmente interessati alle pressioni che ci vengono dall'esterno; se fosse così, non avremmo avuto il coraggio di rischiare spesso la vita in processi pericolosissimi. Certo è - per tutti voi che conoscete bene l'ambiente - che il timore invece sorge rispetto alle ingiustizie che per camarille associative moltissimi magistrati hanno dovuto subire.

Signor Presidente, a poche settimane dalla scadenza del 31 luglio (fino a questo giorno la riforma Castelli è stata sospesa in alcune sue parti dalla legge n. 269 del 2006), la magistratura italiana non solo non ha un nuovo ordinamento giudiziario, ma non sa nemmeno quale sarà la proposta definitiva della maggioranza di Governo. Voci allarmate si susseguono infatti sia nel mondo della magistratura, sia nel mondo dell'avvocatura. I magistrati, almeno per ora, non sciopereranno contro il disegno di legge Mastella, ma la giunta dell'Associazione nazionale magistrati ha deciso ieri di dimettersi. Il parlamentino dell'ANM, dopo ore di discussione, pur giudicando «inaccettabile» il provvedimento licenziato ieri dalla Commissione giustizia del Senato, ha respinto, dividendosi, la proposta di uno sciopero immediato. E ha invece accolto le dimissioni presentate dalla giunta dell'Associazione come gesto di protesta nei confronti della riforma. La questione sciopero però non è definitivamente archiviata: il parlamentino si riunirà nuovamente nei prossimi giorni per discuterne, alla luce dell'*iter* della riforma a Palazzo Madama. La decisione della giunta dell'ANM di dimettersi è un segnale del dissenso della magistratura sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Nella mozione approvata dal parlamentino si esprime, infatti, una valutazione «severamente critica» sul testo licenziato dalla Commissione giustizia del Senato. Su mandato del parlamentino la giunta, pur dimissionaria, continuerà «a seguire con attenzione l'andamento dei lavori parlamentari». Il 10 luglio l'ANM tornerà a riunirsi «per la valutazione delle iniziative da intraprendere, compresa l'eventuale proclamazione di uno sciopero». Alcune parti della magistratura manifestano viva preoccupazione per il fatto che, pur avendo a suo tempo salutato con favore la presentazione del disegno di legge Mastella, senza rinunciare ad evidenziarne i limiti e le criticità, l'impianto originario abbia subito modifiche che sembrano destinate a snaturane l'impronta originaria. La magistratura riconosce come priorità assoluta quella di evitare l'entrata in vigore della controriforma Castelli e comunica anche quali dovranno essere i punti irrinunciabili della riforma che dovrà essere approvata quali consistono nel sistema di valutazioni periodiche di professionalità che deve andare a prendere il posto dell'inaccettabile - secondo loro - meccanismo dei concorsi, nella temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive e nella regolamentazione delle incompatibilità in caso di passaggio di funzioni che non segni nella realtà dei fatti una separazione tra le carriere. Rispetto a questi nodi essenziali, la magistratura non intende accettare nessun regresso e nessun ripensamento e si mostra molto preoccupata per quanto viene riportato sugli articoli di stampa che parlano di snaturamento del disegno di legge Mastella rispetto alla sua impronta originaria. Oggi, di fronte al concreto pericolo di una deriva che la magistratura italiana non può accettare, l'iniziativa dell'ANM è stata ferma e determinata nella sua presa di posizione «per ribadire ancora alla pubblica opinione che i temi della giustizia e dell'indipendenza dei magistrati riguardano da vicino la qualità della democrazia del Paese». E sullo sfondo appare la minaccia dello sciopero. considerare anche la posizione degli avvocati penalisti che manifestano un'adesione quasi totale allo sciopero indetto dall'Unione camere penali italiane contro il disegno di legge Mastella di riforma dell'ordinamento giudiziario. Secondo i dati diffusi due giorni due giorni fa da questa associazione nel corso dell'assemblea nazionale che si è tenuta nella capitale, l'astensione dalle udienze è stata altissima in città come Roma, Milano, Firenze, Napoli e Catania. L'assemblea nazionale, dal tema «In difesa della Costituzione per una riforma democratica e liberale», ha aperto la tre giorni di sciopero. I penalisti, infatti, si sono astenuti dalle udienze fino ad oggi. I primi dati dell'astensione, che si è attestata ben oltre il 90 sono stati resi noti ieri dall'associazione nel corso della manifestazione che si è svolta nella cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. I penalisti hanno spiegato che l'aver «deciso di incrociare le braccia è il segnale di un malessere». Per il presidente delle camere penali «forse la politica della giustizia non ha mai toccato un livello così basso». E ha continuato: «Le modifiche al disegno di legge Mastella definitivamente approvate in Commissione giustizia del Senato suscitano le più ampie critiche, anche per ragioni di metodo». «L'ANM» - ha concluso il presidente - «ha dettato le regole a colpi di minacce di sciopero: sappiamo benissimo che segue questa prassi costante ed insistente, ma non arriva mai a proclamare lo sciopero perché minacciarlo è quanto le basta per ottenere quasi incondizionatamente quello che chiede». Affrontiamo ora il contenuto del provvedimento in discussione. II disegno di legge Mastella non solo riforma in modo deciso il decreto Castelli riguardo agli aspetti coinvolgenti la carriera dei magistrati, ma tocca qua e là anche altri decreti sull'ordinamento giudiziario, e cioè alcune norme già approvate ed entrate in vigore, al dichiarato fine di valorizzare l'aspetto sistematico della normativa. In realtà, la priorità assoluta è rappresentata dalla esigenza di evitare l'entrata in vigore della riforma Castelli, approvata nella scorsa legislatura con fortissime resistenze da parte della sinistra e di certi settori della magistratura, ostili al cambiamento di una legge che risale al lontano 30 gennaio 1941 e che attendeva di essere riformata da oltre cinquant'anni. Alla riforma Castelli va riconosciuto il merito di aver affrontato per la prima volta in modo sistematico una materia così complessa proponendo soluzioni innovative, alcune delle quali hanno dovuto necessariamente venire apprezzate da parte dei maggiori detrattori della riforma, come ad esempio in tema di scuola della magistratura, di consigli giudiziari, di tipizzazione degli illeciti disciplinari che sono stati per la prima volta, appunto, tipizzati. Ricordiamo che nel corso dell'attuale legislatura il Parlamento ha già approvato la legge 24 ottobre 2006, n. 269, che è intervenuta su tre su tre dei decreti legislativi attuativi della riforma, disponendone, secondo i casi, la sospensione dell'efficacia o la modifica del contenuto. In particolare, sono stati cambiati alcuni punti dei decreti relativi all'assetto dell'ufficio del e agli illeciti disciplinari dei magistrati, mentre - appunto - è stata differita l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 160 sull'accesso, la carriera e le funzioni dei magistrati, in quanto il ministro Mastella - e la magistratura - lo ha ritenuto difficilmente emendabile e comunque meritevole di una riforma più articolata e approfondita. Ma il tempo stringe e il Parlamento ha davvero poco tempo per l'approvazione definitiva: se questa non avverrà entro il 31 luglio, rivivrà il decreto Castelli. Inoltre, risulta chiaro a tutti come la materia dell'ordinamento giudiziario sia estremamente delicata perché carica di conseguenze non solo e non tanto per i diretti destinatari della stessa (ovvero i magistrati), quanto piuttosto per gli utenti del servizio pubblico e, più in generale, per la stessa società civile. Porre fine a questo stato di incertezza dovrebbe essere la priorità assoluta del Governo, che ha preferito mettere mano ad una riforma appena varata nella scorsa legislatura, senza, al contempo, garantire la sua approvazione entro i tempi previsti. Il risultato non è di poco conto per la fondamentale importanza che riveste la riforma dell'ordinamento giudiziario, in quanto, tra i fattori che determinano il cattivo funzionamento del sistema giustizia del nostro Paese e la conseguente fuga dalla giurisdizione pubblica, un ruolo fondamentale lo riveste proprio l'inadeguatezza degli ordinamenti e delle regole che servono a plasmare la qualità dei soggetti-protagonisti della giurisdizione, avvocati e magistrati. Esaminando nel dettaglio la riforma Mastella, vediamo come la disciplina del concorso per l'accesso in magistratura tenti di ovviare ad alcune storiche problematiche, già affrontate dalla riforma Castelli, legate in particolare alla lunghezza delle procedure concorsuali e all'inadeguatezza delle prove scritte d'esame, oramai superate per il loro taglio prevalentemente teorico. Purtroppo sono stati eliminati alcuni punti fondamentali e innovativi della riforma precedente, come l'indicazione obbligatoria da parte del candidato dell'area funzionale cui accedere in caso di esito positivo del concorso (giudicante o requirente), e la specifica prova psico-attitudinale da sostenere nelle prove orali. Va sottolineato 1'aspetto critico di questa riforma, ovvero l'aver rinunciato all'obbligo iniziale di scelta definitiva tra funzioni giudicanti e requirenti, che sarebbe servita a porre fine alla continua commistione tra giudici e pubblici ministeri ministeri cui abbiamo spesso assistito, e avrebbe consentito di raggiungere una marcata distinzione tra le due funzioni che avrebbe potuto successivamente portare alla definitiva separazione delle carriere. Riguardo ai requisiti per l'ammissione al concorso, dobbiamo notare come viene confermata la linea ispiratrice della riforma Castelli impostando, seppur con correttivi, il concorso di magistrato ordinario come concorso di secondo grado. Inoltre, la riforma Mastella, pur introducendo rilevanti modifiche alla disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati come prevista dalla riforma Castelli, ha dovuto riconoscere che il sistema di valutazioni di professionalità anteriore alla legge n. 150 del 2005 non era più adeguato perché basato su presunzioni e verifiche limitate, complessivamente insufficiente ad attuare un reale vaglio delle specifiche capacità richieste. La nuova disciplina ha previsto valutazioni di professionalità ogni quattro anni, sganciate dagli scatti di carriera, consentendo così un monitoraggio continuo della professionalità in modo da rendere possibile individuare le sacche di inoperosità, spesso lamentate da parte di alcuni operatori del diritto e che già la riforma Castelli aveva tentato di arginare. Tuttavia, va sottolineato il rischio evidente connesso alla progressione in carriera e alle valutazioni di professionalità, dove il meccanismo rimane tuttora nelle mani della magistratura, con evidente inversione di rotta rispetto alla riforma Castelli che aveva limitato notevolmente il ruolo del CSM. La valutazione si basa su giudizi espressi dai consigli giudiziari e dal Consiglio superiore della magistratura, che sono organi del circuito di governo autonomo e dove i magistrati eletti sono in netta prevalenza; in altri termini, le valutazioni di professionalità continuano ad essere effettuate proprio da chi viene eletto dai soggetti che deve valutare: quindi il controllato elegge il controllore. Di certo va valutata negativamente la riduzione dell'apporto, nella valutazione, di elementi esterni alla magistratura, e in particolare dell'avvocatura, la cui presenza nel progetto Castelli è senz'altro più forte e il cui contributo La riforma Mastella introduce, nell'arco della carriera del magistrato, i concorsi per soli titoli (la riforma Castelli prevedeva anche quelli per esami) a cui può partecipare solo chi abbia superato le richieste valutazioni di professionalità. In ogni caso, sembra che ci si sia resi conto dell'importanza di bandire ogni forma di progressione automatica e di configurare la progressione in carriera unicamente alla luce di profili meritocratici. La progressione economica viene sganciata dalle funzioni, circostanza che dovrebbe costituire un possibile stimolo per magistrati esperti a permanere nelle funzioni di primo grado che tanto interessano i cittadini, perché è quello che le parti conoscono e da cui attendono risposta adeguata e sollecita alla propria domanda di giustizia. Inoltre, viene previsto un meccanismo per cui il magistrato non idoneo viene penalizzato e alla fine anche rimosso; l'idoneità del magistrato viene valutata non solo sulla base delle sue conoscenze tecniche, ma anche sulla base di una serie di altri parametri che costituiscono tutto quel bagaglio di caratteristiche con cui si svolge la funzione, dall'operosità all'equilibrio, all'equilibrio, dalla capacità organizzativa alla preparazione, all'attitudine alla dirigenza. Per quanto riguarda gli incarichi direttivi, sono previste alcune regole già contemplate dalla riforma Castelli e riconosciute oramai come indispensabili, come la temporaneità e il nuovo concorso per l'unico rinnovo possibile dell'incarico; la specifica valutazione della capacità direttiva; la previsione di un meccanismo di controllo sulla gestione da effettuarsi ogni due anni e che può portare anche alla revoca dell'incarico; l'attribuzione di un ruolo di impulso e di gestione, nonché del compito di relazionarsi con gli altri uffici giudiziari, e infine di consultare per il programma annuale anche il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, in un'ottica di condivisione e di partecipazione da valutare positivamente. Si prevede che il magistrato ordinario, dopo il tirocinio, non possa - fino a che non è valutato almeno una volta sotto il profilo dell'equilibrio della competenza, della preparazione, della capacità organizzativa - assumere la funzione di pubblico ministero o GIP singolo, che può decidere sulla libertà personale dei cittadini. In nome della doverosa attenzione alla professionalità del magistrato, la riforma Castelli ha istituito la scuola superore della magistratura, una struttura stabile incaricata di occuparsi in maniera continuativa delle esigenze formative e di aggiornamento per il personale di magistratura e per il tirocinio degli uditori giudiziari senza funzioni. Tale scelta è stata giudicata condivisibile dall'attuale Ministro, soprattutto per quanto riguarda la individuazione di uno strumento preposto alla formazione professionale dei magistrati, sino ad oggi garantita dal CSM. Tuttavia, la riforma Mastella - probabilmente anche a seguito di pressioni - ne ha corretto la impostazione iniziale che vedeva attribuite alla scuola molte funzioni legate alla progressione in carriera ed alla preparazione e svolgimento dei concorsi. Sotto questo aspetto, infatti, il testo Mastella appare frutto di un compromesso che colloca la scuola in un ambito più ristretto, investendola esclusivamente del compito di curare l'attività di formazione iniziale, complementare e permanente dei magistrati, e di riconversione a seguito del passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa. Resta da aggiungere che la lettura dei lavori della Commissione giustizia, soprattutto in riferimento alla decisione di stralciare alcuni articoli del disegno di legge (con un continuo cambiamento su alcuni aspetti rilevanti del provvedimento), induce a ritenere che siamo di fronte ad una inutile controriforma dell'ordinamento giudiziario. Oltre a queste considerazioni, per così dire, istituzionali, ci sarebbero poi da aggiungere una serie di considerazioni che dovrebbero essere basate sull'esperienza di vita quotidiana che tutti i cittadini, compresi noi, credo abbiamo avuto la ventura di vivere. Qui si parla in maniera altisonante, aulica in questa che è la Camera alta del Parlamento di cose di certo estremamente importanti per la vita democratica ma non solo quotidiana del Paese e dei suoi cittadini, ma si dimentica di dire altre cose di assoluto buon senso che ovviamente in queste sedi, siccome non appartengono al politicamente corretto, non vengono mai ricordate. mai ricordate. Se parliamo di necessità di riforma della giustizia, come qualche collega prima ha ricordato, è perché evidentemente il sistema giustizia in Italia non funziona come dovrebbe, altrimenti a nessuno

il doppio o il triplo di Paesi equivalenti al nostro, una cosa comune in tutto quello che è pubblico nel nostro Paese; che la sola Campania ha un numero di magistrati equivalente a quello dell'intera Gran Bretagna; ciononostante, abbiamo 10 milioni di processi civili arretrati *in itinere* e la media della durata dei processi è di quasi dieci anni. Di fronte a queste cose non ho mai sentito un'autocritica dei magistrati, compresi quelli

in tal senso? Credo che a tutti sia capitato, purtroppo, di calcare qualche volta il il suolo dei nostri tribunali e la situazione non può essere sfuggita a nessuno. Anche a me, per varie questioni, ad esempio per le attività amministrative locali che ho svolto per anni, mi è capitato di andare spesso in tribunale per questioni legate a

a cui si era interessati era la quarta o la quinta della mattinata; quindi, c'era il sindaco, il capo dell'ufficio tecnico, il capo dei vigili, eccetera, quattro o cinque persone pagate dai contribuenti, cinque ore ad aspettare il giudice;

ho dovuto partecipare ad una causa di lavoro che dura ormai da quattro o cinque anni e, nonostante le cose che in quest'Aula vengono dette sulla professionalità e quant'altro, il giudice, mentre con gli avvocati ero seduto davanti a lui,

i magistrati eletti mantenevano progressione di carriera e stipendio in aggiunta alla retribuzione da parlamentare? Sono un dirigente d'azienda, ho studiato ingegneria al Politecnico di Milano, ho conseguito un *master* in direzione aziendale, quindi non ho studiato meno di un giudice, forse anche qualche anno di più, ciononostante, quando sono stato eletto, ho dovuto rinunciare al mio posto di lavoro, alla progressione di carriera: il giorno che dovessi ritornare a lavorare dovrò ripartire da zero, nel frattempo non sono maturati gli scatti come per i magistrati. Ecco, di tutte queste cose, e di tante altre di cui si dovrebbe parlare, qui non si parla mai; qui si fanno solo i grandi discorsi teorici che però, ripeto, al popolo non interessano: il popolo vorrebbe avere una giustizia giusta, un magistrato ragionevole che quando ti convoca ti tratta da cittadino suo pari e che in un tempo ragionevolmente breve porta a conclusione i processi, cosa che non avviene in Italia,

Comunque, l'ordinamento giudiziario, pur come un sistema di norme complesso, stratificato, è apparso anche a noi che ci abbiamo lavorato in questi giorni spesso arido, tecnico, amministrativo, una questione per «addetti ai lavori», che può tutt'al più interessare alcuni corpi professionali, come i magistrati, gli avvocati, che viene spesso rappresentata all'opinione pubblica, a chi non fa parte di questi corpi, soltanto come una materia che attiene anche a rapporti di potere tra queste corporazioni e tra la politica e queste corporazioni. Se guardiamo i commenti nelle pagine dei giornali di questi giorni dedicati alla materia di cui ci stiamo occupando questo sembra l'unico interesse, l'unica ragione per scrivere e soffermarsi sul tema dell'ordinamento giudiziario. Certo questo contribuisce a rendere la giustizia e l'organizzazione e il funzionamento della giustizia molto lontani dall'interesse dei cittadini. Non

cosa vuol dire governo delle leggi. Se penso a quanto accaduto ieri su una delle norme più importanti, quella della rappresentanza, ho motivo di dubitare che si abbia chiaro cosa distingue un governo delle leggi dal governo degli uomini, degli esseri umani, e perché le democrazie hanno scelto di ancorare il governo alle leggi. governo alle leggi. Tornando al rapporto tra questa forma di governo, per cui la legge è il limite e la forma dell'esercizio delle funzioni e dei poteri, e la riserva di giurisdizione, vuol dire attribuire a un organo imparziale, indipendente, la funzione e la competenza di valutare e di intervenire sull'applicazione e sul rispetto delle leggi. Il procedimento giudiziario, cioè, è proprio uno dei momenti più delicati ed importanti in cui la legge entra nella vita quotidiana delle persone, nei rapporti concreti tra gli esseri umani umani e vi può entrare fino a limitare la libertà personale, come avviene nel procedimento penale. Quindi c'è un nesso forte, un rapporto stretto tra libertà e giurisdizione che può essere perfino più incisivo

le parole di un filosofo che amo molto, Walter Benjamin, il quale ha scritto in una sua pagina che soltanto il giudice è tra coloro che possono infliggere il destino agli esseri umani perché colpiscono non l'uomo in sé, ma la nuda vita che è in lui. Dunque, chi e come esercita la funzione di amministrare la giustizia deve trovare proprio nell'ordinamento, cioè nel sistema di norme che regola questa amministrazione, le garanzie non per sé, per il magistrato, non per una professione, una corporazione, ma proprio per la funzione che svolge, una funzione che deve essere garantito venga svolta nell'unico vincolo di riferimento alla legge per tutti i cittadini e le cittadine. Quindi, le garanzie che la Costituzione ha posto come princìpi che dovrebbero guidare la costruzione, l'organizzazione, quello che chiamiamo l'ordinamento giudiziario, quei princìpi di indipendenza e di imparzialità, di autogoverno della magistratura non sono prerogative di un potere o di un corpo dello Stato, bensì garanzie per la giustizia e quindi per noi tutti, a partire da quelle di cui si occupa questo disegno di legge, ossia quella della professionalità, della formazione, della valutazione, dell'organizzazione degli uffici, della direzione, della separazione delle funzioni, per stare agli aspetti più rilevanti del disegno di legge in esame. Voglio richiamare come l'elemento dell'indipendenza e dell'autonomia che più direttamente attiene alle

dai poteri, dalla struttura gerarchica e verticale dell'amministrazione della giustizia. Ebbene, il ripristino di una gerarchia e di poteri verticali è stata una delle caratteristiche della della riforma Castelli, cioè di quel disegno di riforma dell'ordinamento su cui l'attuale proposta di disegno di legge approvata in Commissione interviene con rilevanti segni di discontinuità.

precedente, quello costruito nel corso del tempo. L'ultimo intervento legislativo rilevante fu quello di Grandi nel 1941, rispetto al quale gli interventi successivi non sono stati organici e sistematici; è quindi creata una discrasia tra l'ordinamento, sia pur corretto con interventi delle sentenze della Corte costituzionale oltre che di modifiche legislative, e i princìpi stessi della Costituzione, quei princìpi che furono ispirati a una valutazione dell'importanza dell'indipendenza dei giudici proprio dalla struttura gerarchica, dal potere dei vertici che possono limitarla. Era un principio caro a Piero Calamandrei, che ha segnalato proprio il rischio che l'indipendenza restasse una mera idealità se non veniva tradotta in una organizzazione che ridimensionasse il ruolo dei dirigenti degli uffici e mettesse i magistrati tutti sullo stesso piano, creando soltanto una distinzione delle funzioni che esercitano. È a questo criterio che l'attuale disegno di legge si è ispirato ed è su questo che ha segnato una discontinuità. Anche a questo criterio era orientata la scelta che il costituente ha fatto di prevedere un organo dell'autogoverno e anche qui, nell'intervento operato con l'attuale disegno di legge rispetto alle alle modifiche introdotte dalla riforma Castelli, si sono volute riattribuire al Consiglio superiore della magistratura competenze e funzioni che erano state pesantemente ridimensionate e ridotte; ma

Di Lello Finuoli ha definito una «giurisdizione domestica», una funzione troppo interna, che spesso nella prassi ha orientato il funzionamento del Consiglio.

con la riforma Castelli, e però di fare proprie le esigenze di una riforma organica. La discontinuità sta proprio nel fatto che si è cercato di rendere più forti, più espliciti, più chiari i nessi tra i princìpi costituzionali e l'effettivo funzionamento del sistema giudiziario. I punti più qualificanti, infatti, sono quelli che stabiliscono una distinzione netta delle funzioni, rigorosamente definita nei tempi, nei modi e negli effetti. Credo vada sottolineato che la distinzione delle funzioni, quanto agli effetti, cioè il cambiamento dei distretti (il magistrato che cambia funzione non può esercitarla nello stesso distretto né nella Regione, ove la Regione comprenda più distretti giudiziari), opera anche sui dirigenti, cioè su

altri. È proprio rispetto a queste funzioni e alle responsabilità che esercitano rispetto all'organizzazione tutta della magistratura che i cittadini devono trovare una garanzia dell'imparzialità e dell'indipendenza e dell'assenza di confusioni di ruoli del non

modifiche rilevanti rispetto alla riforma Castelli è quello dei Consigli giudiziari e del rapporto con l'avvocatura, cioè della presenza dentro queste strutture degli avvocati, o comunque di soggetti estranei alla magistratura. Si tratta di un'apertura importante per coinvolgere nelle funzioni di valutazione

anche se ovviamente l'avvocato è la controparte nel processo, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, bisognerebbe invece arrivare ad un coinvolgimento che renda possibile la valutazione sull'operato del magistrato anche di chi ne vede la funzione svolta da un punto di vista di parte, che poi è la parte del cittadino. Il terzo aspetto importante è proprio quello dell'accesso, uno degli elementi di discontinuità più rilevanti con la riforma Castelli, che aveva introdotto appunto il «concorsificio», la carriera della magistratura fin dai primi gradi. Io non sottovaluterei una serie di innovazioni che abbiamo introdotto (ne parlava il senatore D'Ambrosio), a partire da quella per cui si tratta di un concorso di secondo grado; ma anche la garanzia, per ai giudici di prima nomina, di cominciare da subito l'esperienza della loro funzione nella collegialità, nel coinvolgimento con gli altri magistrati che hanno un'altra esperienza, perché sono già introdotti nella professione prima di loro; e, nello stesso tempo, equilibrare questa funzione e questa collegialità con un'apertura che viene offerta ai giovani magistrati di poter acquisire posizioni di responsabilità - parlo della quota di riserva per i concorsi anche prima di aver superato i gradi successivi di valutazione. Mi sembra importante che nel disegno di legge vengano definiti i parametri per la valutazione di professionalità:

Certo, si tratta di vedere nella prassi come funzionerà il giudizio, come opererà il Consiglio superiore della magistratura e come opereranno i Consigli giudiziari. Tutto ciò sta anche a noi, sta anche a noi, ma dipende altresì da come le norme scritte in questo disegno di legge, se approvate, contribuiscono o meno a modificare la cultura e la pratica della loro applicazione. Concludo

e tra maggioranza e opposizione. La maggioranza si è ritrovata coesa intorno a questo testo e nel confronto con il Governo (ringrazio tra l'altro il sottosegretario Scotti per il modo con cui ha partecipato e contribuito ai lavori della Commissione),

L'opposizione, pur avendo partecipato con impegno ai lavori, nel giudizio conclusivo ha confermato la sua contrarietà sui suoi punti qualificanti

Abbiamo avuto un confronto libero, come era giusto e doveroso che fosse, che si è espresso in un giudizio finale favorevole a questo testo; ritengo dunque che tale giudizio impegni la maggioranza all'approvazione di questo testo.